Comunico che in data 19 luglio 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69,

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori partendo da una notizia di cronaca di questi giorni, riportata dal quotidiano "La Repubblica" domenica,

Vive da recluso perché è al seguito dei genitori, che sono stati condannati e sono reclusi appunto a Rebibbia. Io penso, noi pensiamo, che nel 2024 sia intollerabile che ci siano ancora dei bambini costretti a scontare la pena dei genitori

di cui sette proprio in istituti penitenziari. Sono bambini che vivono dietro le sbarre e la cui vita è condizionata e sarà condizionata pesantemente da questa loro situazione, di cui ovviamente non hanno colpa. Ora noi pensiamo che su questo tema occorra fare qualcosa. Non è accettabile né tollerabile che ci siano ancora bambini che, in violazione delle Convenzioni, anche della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, sono costretti a scontare la pena dei loro genitori. Chiediamo che su questo sia resa una informativa urgente da parte del Ministro della giustizia

delle detenute madri che consentissero di superare il problema. Mi faccia dire anche, signor Presidente, che sul tema delle carceri c'è un modo di procedere che pensiamo sia altrettanto inaccettabile: stiamo discutendo e inizieremo tra poche ore la discussione sugli emendamenti al decreto-legge sulle carceri, che è composto di 13 articoli. Ebbene, tra ieri sera e stamattina, dai relatori e dal Governo sono arrivati emendamenti che introducono ulteriori 14 articoli. su un decreto di 13 articoli, emendamenti dell'ultimo minuto introducono 14 nuovi articoli. *(Applausi)*. Come si fa a lavorare in queste condizioni? È impossibile. Non è accettabile che si affronti un tema come quello delle carceri, che è nell'agenda delle emergenze di questo Paese, in un modo del tutto confuso e disomogeneo. Crediamo, Crediamo, a questo punto, che anche sul tema affrontato nel decreto carceri, che meriterebbe ben altra attenzione e ben altra organizzazione da parte del Governo, forse sarebbe il caso che la maggioranza si fermasse,

cento delle carceri prevede meno di tre metri quadrati a persona. Signora Presidente, diamo meno spazio ai detenuti di quanto ne diamo ai suini nelle porcilaie degli allevamenti del nostro Paese, con tutto il rispetto per i suini e per l'industria

abbiamo ascoltato degli esperti, abbiamo scritto gli emendamenti sulla base di quelle audizioni. E stamattina ci arrivano 15 emendamenti su un decreto-legge di 13 articoli e noi dovremmo approvarli così.

diciamo alla ministra Alberti Casellati che c'è una riforma che può rendere molto più efficace e molto più allineati alle volontà del Governo, che è quella di chiudere il Parlamento. Se l'Esecutivo emana i decreti-legge, ci fa lavorare su un decreto-legge, dopodiché ci manda gli emendamenti stamattina e fissa il termine per i subemendamenti alle ore 14, poi mette la fiducia su un decreto-legge che va convertito entro il 2 settembre - per cui c'è anche la pausa estiva - che verrà mandato alla Camera per una lettura di

accade in tema di giustizia, cioè sullo *status libertatis* dei cittadini. In quel decreto-legge c'è un nuovo reato - è già legge dello Stato perché quello è un decreto-legge e oggi il Governo che ha scritto quel reato lo modifica quando è già nella realtà, è già nell'ordinamento giuridico. Quindi andiamo a cambiare un reato che è già in vigore. Immagini che i giudici dovranno applicare queste varie leggi che si succedono nel tempo, contraddicendosi l'una con l'altra. Io credo che in democrazia, signora Presidente, le forme siano sostanza. In questo caso si sta svuotando il meccanismo della democrazia parlamentare ed è inaccettabile. *(Applausi)*. Presidente, io vorrei suo tramite far presente che questa maggioranza e questo Governo sono pericolosi: ma non solo pericolosi, sono fascisti, perché i loro metodi sono fascisti.

che ciascuno di voi - cari colleghi della maggioranza - trascorresse almeno quarantott'ore della sua vita in una qualsiasi delle nostre carceri, e poi ne riparliamo. I numeri parlano chiari: 58 morti per suicidio ad oggi nelle nostre carceri. Si tratta di una enormità: equivale a dire a un suicidio ogni tre giorni, a a cui vanno aggiunti anche i sei agenti che hanno deciso di togliersi la vita. Il ministro Nordio ha tanto a cuore questo problema e quindi annuncia da mesi un decreto svuota carceri. Fatalità, signora Presidente, nel frattempo il decreto-legge cambia nome e prende quello di carceri sicure.

luogo, per la mia storia personale, e con tanti difetti, io non posso accettare accuse di estremismi di destra o di sinistra e soprattutto le rimando al mittente. Tuttavia, vorrei occuparmi un attimo solo della mia storia tecnica: neuropsichiatra, sempre dalla parte del bambino, con qualche difetto, ho denunciato da sempre i problemi del sovraffollamento carcerario, dando per acquisito che il sistema della giustizia sia sano,

nella nuova edilizia carceraria, accusandoci di essere medievali e oscurantisti. Rimando al mittente questa accusa, vergognandomi un po' per lui.

presenza in Aula, ero tra coloro che disturbavano durante gli interventi. Poi ho capito che è molto meglio ascoltare quello che l'opposizione dice, per poi ribattere. Magari anche loro prenderanno la parola dopo e potranno ribattere, ma che ora ascoltino in serenità come ha fatto la maggioranza. Detto questo, la situazione carceri che abbiamo trovato è talmente drammatica che, a venti mesi dall'inizio del mandato del Governo Meloni, abbiamo iniziato a metterci mano. metterci mano. Questo non significa fare quello che le opposizioni non hanno fatto nei precedenti dieci anni. con i genitori che hanno commesso dei reati non perché il Governo Meloni si è svegliato e ha deciso di incarcerare i genitori; padre e madre hanno commesso dei reati e sono stati puniti. Sul fatto che non ci sia ad oggi - questo grazie a voi - uno strumento che consenta un'altra possibilità per quel bambino, sinceramente mi farei una domanda. *(Applausi)*. Il sistema *(Applausi)*. Il sistema carcerario è un mondo talmente delicato e particolare che, se credessimo davvero tutti al recupero del detenuto che ha commesso un grave errore, non staremmo qua a tirarci i capelli

recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca"

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 1.193, d'iniziativa del Governo, appena licenziato dalla 7a Commissione nella seduta odierna, nel medesimo testo approvato dalla Camera in prima lettura. Il provvedimento è suddiviso in quattro capi. Il capo I, dall'articolo 1 all'articolo 5, reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e sulla relativa disciplina fiscale. L'intervento legislativo risponde innanzitutto alla necessità e urgenza di fornire sostegno sia agli organismi di enti sportivi, mediante disposizioni volte a rendere maggiormente qualificate le elezioni dei loro componenti, e a introdurre l'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni, sia anche all'associazionismo di base, in attuazione di quanto è previsto dall'articolo 33 della Costituzione, nonché in considerazione dei valori educativi, sociali, di sviluppo e di benessere psicofisico connessi all'attività sportiva. Ulteriori disposizioni concernenti le prestazioni di lavoro sportivo si inseriscono nel processo in atto di affinamento della normativa in materia di lavoro nello sport (alla luce anche della verifica dell'impatto della stessa), promesso da questo Governo al momento dell'insediamento. Ricordate che il provvedimento era del Governo precedente. Al riguardo, segnalo che alcune disposizioni del presente decreto sono in linea con alcune specifiche indicazioni che stanno emergendo in sede di esame da parte della Commissione cultura e sport del Senato sull'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio (Atto n. 373). Nel capo II, articoli dal 6 al 9-*bis*, si introducono disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità. disposizioni muovono dalla necessità, ormai improcrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati nel sostegno didattico agli alunni con disabilità. A favore delle persone con disabilità si dispone un incremento del relativo fondo, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, inserendo fra le sue finalità il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia nelle scuole secondarie di secondo grado. Altre disposizioni rispondono alla necessità di ridurre l'ingente mole di istanze già presentate al Ministero dell'istruzione al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito all'estero per lo svolgimento di attività didattiche rivolte agli alunni con disabilità. Si procede altresì al riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), al quale è affidata anche l'attivazione di specifici percorsi formativi per il sostegno agli alunni con disabilità. Il capo III, articoli dal 10 al 14-*quater*, detta disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025. Tali disposizioni incidono sia sul reclutamento del personale docente, sia sul sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Si interviene inoltre per promuovere una compiuta accoglienza e integrazione scolastica degli alunni stranieri. Il capo IV, articoli dal 15 al 17, reca disposizioni urgenti in materia di università e di ricerca, in attesa dell'approvazione di una riforma per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione del cosiddetto pre-ruolo universitario e della ricerca. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati accolti dal Governo atti di indirizzo che lo impegnano a valutare l'opportunità di promuovere, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e presso il Comitato italiano paralimpico, azioni di sensibilizzazione per la modifica degli statuti degli organismi sportivi, allo scopo di garantire, con riferimento alla loro disciplina elettorale, una piena partecipazione democratica, attraverso il voto anche elettronico, nonché mediante il rispetto della *governance*, del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di coloro che non abbiano compiuto trentasei

disposizioni in materia di università e ricerca. Siamo evidentemente di fronte all'ennesimo decreto *pot-pourri*.

non risponda ai necessari profili di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della nostra Costituzione, che questa maggioranza sta tentando in ogni modo di mandare in soffitta. Le modalità di adozione del decreto-legge, come i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare, precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina sistematica e meditata di materie

uno strumento non più straordinario, ma ordinario, anzi l'unico strumento con cui si legifera. Eppure la Corte costituzionale si è espressa più e più volte, sottolineando come la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità

Lo stesso Presidente della Repubblica ha censurato questo utilizzo perché è una prassi che continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione

Tuttavia, si procede nella stessa maniera. Come dicevo, questo decreto-legge, in particolare, è caratterizzato anche da un elevato tasso di eterogeneità delle materie trattate. essere di fronte a una serie di norme assemblate insieme più per una casualità temporale, che per un'effettiva loro omogeneità. Passando alle criticità di merito,

che negli organismi delle federazioni sportive debba essere data adeguata rappresentatività alle leghe sportive professionistiche secondo parametri direttamente proporzionali, quindi guardando solo al peso del contributo economico e senza tener conto del numero degli iscritti e dei risultati sportivi e relegando in secondo piano il settore dello sport dilettantistico che tanto ruolo ha nella definizione degli aspetti sociali e di emancipazione, in piena violazione della modifica dell'articolo 33 che tutti insieme, qui dentro, abbiamo votato solo pochi mesi fa. Con riferimento all'articolo 2, si istituisce la commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. - udite, udite - vengono però nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che, quindi, indipendente non è affatto. Appare pertanto decisamente eccessiva l'ingerenza del Governo e della politica nelle norme di un organismo che, per paradosso, viene definito indipendente. *(Applausi)*. Occorre rammentare, poi, come l'articolo 33 della Costituzione l'ho detto poc'anzi - è stato modificato proprio da noi pochi mesi fa per affermare il valore dello sport. È paradossale, pertanto, che a distanza di poco tempo si converta un decreto che ne decreta assolutamente la dipendenza dalla politica.

devono eliminare la richiesta di riconoscimento e fare un percorso di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di un trucco ai danni dei nostri connazionali che hanno legittimamente conseguito un titolo all'estero. Ma c'è molto di più. Ciò è evidentemente frutto dell'incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione adeguata, legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli conseguiti all'estero.

2024 e 2025. Per cosa i contribuenti spendono questi soldi, visto che i riconoscimenti non vengono fatti? Anzi, si chiede ai ricorrenti di togliere ed eliminare la loro richiesta di riconoscimento e fare un percorso di specializzazione, sono soldi buttati assolutamente nel nulla, perché si preferisce ricorrere a un *escamotage*, che peraltro nulla ha a che fare col merito, che pure avete inserito nel titolo di un Ministero. All'articolo 15, infine, altrettanto rilevante è notare la violazione dei diritti di altre categorie estremamente importanti per il nostro Paese: coloro che si dedicano all'attività della ricerca subiscono un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca. Soltanto nel 2022 si era stabilito che si passasse dagli assegni di ricerca ai contratti di ricerca. Ebbene, questa maggioranza, invece, con proroghe continue, continua a tenere la categoria dei ricercatori in uno stato di precarietà. Sono stati introdotti i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni per consentire di passare da un contratto parasubordinato a un contratto determinato di minimo due anni, con maggiori tutele, migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, ferie retribuite e indennità, insomma tutele. Questa maggioranza invece va ancora in proroga e continua a danno dei nostri ricercatori con gli assegni, quindi senza tutele. Appare pertanto ingiustificabile il perenne rinvio di questa disposizione e per tutto quanto detto sin qui, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1193.

disabili non hanno gli insegnanti di sostegno e gli educatori non sono formati in modo adeguato. Queste sarebbero le questioni da discutere e da affrontare, non con urgenza, ma in modo strutturale; invece, siamo sempre di fronte

nostro esame rappresenta un passo fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Esso introduce infatti norme specifiche per migliorare la trasparenza e la gestione delle attività sportive, come il riconoscimento giuridico e l'indipendenza operativa della Nado. Si tratta di passi cruciali per garantire l'integrità dello sport e prevenire fenomeni di corruzione e di *doping*. prevede la proroga necessaria per completare la riforma dei contratti di ricerca, che è fondamentale per attrarre e mantenere i giovani talenti nel nostro sistema accademico. Il raddoppiamento del fondo per i contributi agli affitti per gli studenti fuori sede è una misura concreta che risponde alle difficoltà economiche di molte famiglie, promuovendo anche la mobilità studentesca e l'accesso all'istruzione superiore. Questo intervento non solo allevia il peso finanziario, ma contribuisce a creare una società più equa e dinamica. Per queste ragioni noi rigettiamo fermamente la questione pregiudiziale e ribadiamo il nostro sostegno al provvedimento. *(PD-IDP)*. Signor Ministro, chiaramente lei oggi qui rappresenta il Governo insieme al ministro Ciriani e rappresenta anche uno

la Ministra dell'università e della ricerca. Quando ci si trova di fronte ad un decreto *omnibus* è difficile riuscire a fare un ragionamento organico e provare a spiegare

eravamo illusi per il titolo che reca «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca». Stando al titolo si dovrebbe essere d'accordo. In realtà, però, andando a vedere il contenuto di questo mega contenitore, i motivi che ci portano a dire che non dovrebbe neppure essere affrontato sono tanti. Parto dallo sport; mi dispiace non vedere in Aula il ministro Abodi, che è stato presente in Commissione fino a poco fa e queste osservazioni le abbiamo fatte anche a lui. Mi dispiace perché questo provvedimento per quanto riguarda le misure relative è entrato a gamba tesa - uso questa metafora - rispetto ad un lavoro che questo ramo del Parlamento stava facendo seriamente sul mondo del calcio. Nella 7a Commissione da mesi c'è un affare assegnato sulla situazione del mondo del calcio in modo particolare, affrontato seriamente e trasversalmente

per fare della buona politica. Noi, Ministro, lo dico a lei che se ne farà portavoce con il Governo, abbiamo presentato per l'Aula anche un ordine del giorno che chiede che i risultati di quell'affare assegnato, che è un'indagine conoscitiva molto ricca e approfondita, possano essere utilizzati come base per una riforma più completa di tutto il settore del calcio. *(Applausi)*. Dico

costruito dal Parlamento, che possa parlare a tutti i mondi e che ricordi che cos'è il calcio, che è fatto di professionisti, di allenatori e di calciatori ed è fatto da quei tifosi che vanno allo stadio, che fanno gli abbonamenti, che pagano le *Pay* TV per poter vedere la loro squadra del cuore; è fatto d'affetto, di calore e di passione e ha bisogno di essere affrontato con grande trasversalità. Per questo motivo, la scelta che voi avete fatto, di entrare a gamba tesa e di creare questa sorta di super organismo nominato dalla politica, ci vede profondamente contrari nel merito, ma anche nel metodo Ministro, vado avanti per descrivere cosa c'è in questo provvedimento di altrettanto sbagliato. Mi dispiace doverlo dire, perché rispetto al tema del sostegno il Partito Democratico non ha posizioni ideologiche. Noi sappiamo che la la mancanza di insegnanti di sostegno non è un problema creato da questo Governo. È un problema che noi abbiamo da tantissimo tempo, perché mancano gli insegnanti specializzati sul sostegno. Quindi, siamo assolutamente favorevoli a lavorare insieme per trovare delle soluzioni. Ma le soluzioni che noi riteniamo più corrette vedono una formazione degli insegnanti di sostegno omogenea, non con percorsi di serie A e percorsi di serie B. quello che purtroppo è venuto a mancare in questo provvedimento è affrontare la formazione degli insegnanti di sostegno nel modo più logico possibile,

Quei bambini e quelle bambine che entrano a scuola con un insegnante di sostegno non sono in deroga. Ci sono e rimangono per tutto il loro percorso. Quindi, abbiamo bisogno di questo. Voi, invece di potenziare il grande piano

che noi non condividiamo la vostra scelta, ma, se avete deciso di fare in questo modo, bisognava fare in modo che la macchina dell'INDIRE venisse messa nella condizione di essere oliata e di lavorare nella modalità migliore possibile. Togliete la serenità anche all'INDIRE, commissariandolo, e quindi annullate il ruolo della Presidente dell'INDIRE

sono sicuramente sbagliati, perché il merito non interessa. Mi dispiace, signor Ministro, perché l'altra illusione che voi ci avete dato è quella che vi sareste presi a cuore davvero, visto che la sbandierate in tutto e per tutto, la questione del merito.

se lei fa qualcosa di buono per la scuola, il Partito Democratico glielo riconosce. Lei sa che ci sono delle sedi vacanti, sa che c'è bisogno di avere del personale, dei dirigenti scolastici che siano di ruolo e quindi cerca delle soluzioni. Il problema è che ha cercato una soluzione, accogliendo quell'emendamento, che penalizza i dirigenti scolastici che hanno superato la prova del 2023 e che si troveranno ora, per quell'emendamento che voi, senza nessuna forma di merito, avete deciso di appoggiare, scavalcati da chi aveva perso il concorso del 2017, non lo aveva passato e si trova a fare, attraverso contenziosi, un percorso a parte, avvantaggiato. Andranno avanti rispetto a chi oggi si ritrova a non poter chiudere il

perché anche per quanto riguarda gli alunni stranieri abbiamo tante perplessità. Avremmo voluto che finalmente venisse messo in atto un meccanismo per attuare la vera certificazione linguistica dei ragazzi con *background* migratorio o dei nuovi arrivati in Italia, perché io che vengo da Pioltello, una zona che lei conosce molto bene, conosco benissimo la situazione, come la conosce dei ragazzi che hanno *background* migratorio ma che sono nati in Italia, che frequentano da sempre le nostre scuole, che parlano benissimo l'italiano ma che hanno bisogno di altro per potersi inserire bene, perché vivono male

a fronte di prezzi che giustamente - non stiamo a sindacare questo - aumenteranno. Signor Ministro, lei aveva promesso a settembre dell'anno scorso che avrebbe dato una mano alle famiglie in difficoltà a cominciare l'anno scolastico. Per fare questo, deve fare in modo che la proposta di legge del Partito Democratico sulla gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo diventi la normalità, diventi la legge con cui affrontate la legge di bilancio. *(Applausi)*. Di milioni ne servono 500, tolti 103 sono circa 400, ma è in quel modo che voi andrete incontro alle famiglie che altrimenti a settembre si troveranno a spendere 400 euro per ogni bambino o ragazzo che va a scuola e con i chiari di luna che ci sono non mi sembra che questa sia una buona azione rispetto al diritto allo studio. C'era, infine, un'altra opportunità:

agli enti locali, ma anche a tutti coloro che si occupano di educazione di quella fascia di poter aprire i servizi. Come Partito Democratico abbiamo presentato una risoluzione in Commissione, se voi non aveste, come sempre, la fretta di approvare un provvedimento solo in un ramo del Parlamento non utilizzando l'altro, qui avreste avuto il veicolo adatto per risolvere un problema che trasversalmente vi viene posto. Iniziamo a pensare che esistono due rami del Parlamento, facciamoli lavorare entrambi e non facciamo fare ad un ramo il passacarte dell'altro.

intanto, perché sul tema dello sport finalmente, dopo decenni di silenzio politico, c'è qualcuno come il ministro Abodi che viene, presenzia ai lavori della Commissione, ascolta quanto i parlamentari, in questo caso i senatori, hanno da dire e prende gli aspetti necessari ed urgenti inserirli all'interno di un decreto. Questo fa la differenza e non è un caso che lo sport sia entrato in Costituzione anche grazie all'attività di questa maggioranza; non è un caso che di sport finalmente si torni a parlare. in esame reca la modifica delle prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il riconoscimento del rimborso forfettario per i volontari nello sport;

la continuità dei docenti a tempo determinato sul posto di sostegno, con cui si promuovono i diritti degli alunni con disabilità, non è un aspetto necessario e urgente che noi riconosciamo nelle nostre scuole? La possibilità di avvalersi di esperti per le attività formative a favore di persone con disabilità è davvero così poco importante? Non è davvero necessario ed urgente immettere nel ruolo, con riserva presso le istituzioni scolastiche, tutte le persone che hanno superato il concorso del 2016? Quanti anni dobbiamo ancora aspettare? Non è necessario e urgente? Ci sono poi i soggetti che devono invece rimanere in ruolo e che hanno superato il concorso del 2020: non è necessario e urgente neanche questo? Ci sono i docenti, anzi c'è il docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri, soprattutto per coloro che hanno il primo anno di attività nelle scuole in Italia: non è necessario e urgente neanche questo? Vogliamo abbandonare i ragazzi senza dar loro una vera struttura di sostegno all'inizio dell'anno scolastico? C'è la mobilità interregionale da garantire per l'anno scolastico 2024-2025: non è necessario e urgente neanche questo? C'è da attivare la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici: è qualcosa che vogliamo fare e che rivendichiamo proprio perché siamo il Governo del merito e anche su questo vogliamo fare le nostre valutazioni come è giusto che sia, ed è necessario e urgente farlo prima che inizi l'anno scolastico, o comunque in concomitanza con l'anno scolastico. C'è da assegnare l'incremento di 3 milioni di euro per il *welfare* studentesco e questo è necessario e quanto mai urgente. C'è il contributo per le spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede e anche questo è molto necessario e urgente. Soprattutto, però, ci sono 136.000 alunni con disabilità che al momento non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati sul sostegno.

una serie di contrapposizioni, ricorsi e fattispecie in generale, che finalmente viene risolta con un decreto-legge, perché finalmente diamo la possibilità dall'inizio dell'anno di riconoscere i titoli, i meriti e le qualifiche che questi docenti hanno acquisito. Questo è necessario e urgente. scolastici con una norma di buonsenso, proprio per garantire l'inizio dell'anno scolastico. Siamo a luglio e quindi a settembre questo va garantito: è necessario e urgente anche questo. Soprattutto è necessario e urgente avere la capacità

prima di dichiarare aperta la discussione generale, devo comunicarvi che la Presidenza ha verificato il contenuto dell'intervento della senatrice Cucchi devo segnalare che le parole usate non sono appropriate. *(Applausi)*. Pertanto, colleghi, la Presidenza invita tutti i senatori ad usare un linguaggio che non sia offensivo verso i colleghi. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà. Senatore, poiché la senatrice Malpezzi ha rinunciato al suo intervento, lei ha a disposizione dieci minuti.

che parla di università e racconta molto del modo di fare del Governo della destra. Questa norma proroga fino al 31 dicembre la tipologia dell'assegno di ricerca, che sarebbe dovuta cessare a luglio; una proroga che si aggiunge a una proroga precedente, poi a un'altra ancora e così all'infinito. Che cos'è l'assegno di ricerca? È la fattispecie introdotta nel 2010 da un altro Governo di destra, di cui l'attuale presidente del Consiglio Meloni faceva parte, non come passante ma ricoprendo il ruolo di Ministra. È la tipologia precaria e precarizzante, la tipologia cardine quasi esclusiva del cosiddetto pre-ruolo, ovvero di quel tempo che intercorre per tantissimi giovani ricercatrici e ricercatori tra la laurea, il dottorato e il lavoro a tempo indeterminato. Per oltre il 90 di questi giovani, dopo un precariato che mediamente dura molto più di dieci anni, l'assunzione in ruolo non arriverà mai e non per incapacità o inadempienze, ma per la natura stessa del nostro sistema universitario, fondato fondato strutturalmente sul precariato, sullo sfruttamento del lavoro precario. Di tutto ciò l'assegno di ricerca è il simbolo; il simbolo; il simbolo in tutti questi anni, dello sfruttamento di intere generazioni di talenti, di ingegni, di studio, di passione scientifica. Altro che merito! Altro che meritocrazia! *(Applausi)*. Parole vuote, inganno vostro per i *talk show*, per i salotti della campagna elettorale. In Italia, chi non può permettersi almeno dieci anni di precariato viene espulso dalla carriera universitaria: masticato, utilizzato e poi espulso. La colpa non è del destino cinico e baro, signori del Governo, ma di un sistema cinico e baro che voi state alimentando. Presidente, con migliaia di ricercatori, nelle assemblee e nelle audizioni in Parlamento, noi a questo sistema abbiamo detto di no, con i fatti. fatti. Non si può accettare una incertezza che impedisce di fare ricerca, che mortifica la possibilità di costruire una vita. Abbiamo detto no e questa consapevolezza è nata incontrando ricercatrici e ricercatori, ascoltando una frustrazione collettiva che non è e non può essere considerata un fatto privato, ma è una questione politica primaria e urgente. nell'idea che si ha dell'università, c'è l'idea che si ha del Paese; per questo abbiamo bisogno di un'università che sia più larga e che non sia solo per pochi, ma che sia per tutti, per tutti coloro che vogliono studiare e che oggi sono impediti a farlo. Presidente, non è vero che la politica è tutta uguale. No, non è vero. *(Applausi)*.L'università italiana non si è mai ripresa dai tagli del Governo della destra del 2009-2010: un miliardo e mezzo di tagli, che hanno impedito ad intere generazioni, ragazze e ragazzi delle famiglie meno abbienti, di andare avanti, di credere in se stessi, di realizzare il proprio progetto di vita, di continuare a studiare. Quei tagli della destra sono stati voluti e sono il frutto avvelenato di un'idea sbagliata e classista di società. Non è vero che la laurea non conta, questa è una grande bugia reazionaria. La laurea protegge dalla disoccupazione e dalla marginalità. Studiare conviene sempre; e se potrà essere indifferente per chi vive in una famiglia agiata e ricca, per chi vive in una famiglia povera,

Ecco, Presidente, noi rivendichiamo il fatto che dal 2016 si è riavviata, tra mille difficoltà, una politica di investimenti nell'università, nella ricerca e nel diritto allo studio, con nuovi piani di reclutamento e di assunzioni, dopo gli anni del feroce blocco del *turnover* imposto dalla destra. E rivendico, Presidente, di aver noi qui in Senato condotto, nella scorsa legislatura, un'indagine conoscitiva parlamentare sulla condizione studentesca e sul precariato nella ricerca, perché queste sono le due questioni essenziali di una più grande questione universitaria, che è un grande tema politico che questo Governo continua a rimuovere. Il risultato di quell'indagine ha individuato nell'assegno di ricerca, che noi abbiamo cancellato e che voi prorogate all'infinito, il motivo di un'insostenibile bolla di precariato: cioè nella mancanza del riconoscimento giuridico - e politico - del lavoro della ricerca. Fare ricerca è un lavoro! E come tale va sostenuto e va protetto. Abbiamo bisogno di incentivare una cosa che in Italia è praticamente scomparsa: la ricerca di base, capace di sperimentare sulle frontiere più innovative, così essenziali nel tempo che viviamo della rivoluzione tecnologica, capace di essere coraggiosa, autonoma e indipendente. È per questo, per tutti questi motivi, che nel giugno di due anni fa, dopo una battaglia parlamentare, politica e culturale, abbiamo cancellato l'assegno e introdotto una nuova forma: il contratto di ricerca, lavoro non più precario e molto meglio pagato, comprensivo di tutte le tutele previdenziali e contributive. Parallelamente abbiamo introdotto la figura di ricercatore in *tenure track*, secondo gli standard europei. Abbiamo costruito, per la prima volta dopo il 2010, una vera riforma, nell'interesse non di una parte, ma del futuro e delle potenzialità del nostro Paese. Certo, Presidente, non una riforma perfetta; però una riforma con una visione, con un'idea avanzata ed espansiva di università e di società. Il Governo Meloni, in questi due anni, ha impedito in ogni modo l'attuazione di questa riforma, non finanziandola e

con l'introduzione di una nuova selva di contrattini ultra-leggeri, ultra-precari, malpagati e senza diritti, che allungheranno il precariato fino alla soglia della e che renderanno il nostro sistema meno attrattivo e meno competitivo. Altro che fandonie! I nostri laureati vanno all'estero perché il nostro sistema è nuovi tagli all'università, come quelli denunciati qualche giorno fa dai rettori; oltre 500 milioni di tagli al fondo ordinario che mettono a rischio la sopravvivenza stessa del sistema delle università pubbliche e lo disgregano. Altri tagli lineari si annunciano in legge di di bilancio. Presidente, con la fine dei fondi del PNRR molti atenei più piccoli saranno costretti a un nuovo blocco del *turnover*, forzosamente, e molti altri rischiano il dissesto e la chiusura, con il rischio di desertificazione di interi territori. In questo decreto la destra toglie soldi al reclutamento per metterli sulla progressione delle carriere. Si tratta di un cortocircuito pazzesco, inaccettabile. Servono investimenti per gli uni e per gli altri, non gli uni contro gli altri. Concludo, signor Presidente. In questi giorni, dopo due anni, si svela l'idea di università della destra: il definanziamento e l'attacco ai diritti appena conquistati dai lavoratori della ricerca. Così facendo, il Governo Meloni fa pagare la crisi al precariato universitario e ai ragazzi più giovani, per i quali sarà sempre più difficile mantenersi agli studi e pagare una stanza, i libri, una mensa.

sia un Governo che, in due anni, non ha dato alcuna risposta agli studenti in tenda, sfrattati a causa di affitti insostenibili;

Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, questo disegno di legge comprende 17 articoli che investono 4 ambiti: sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di ricerca e università e misure urgenti per promuovere il regolare avvio dell'anno scolastico. In Commissione abbiamo presentato 117 emendamenti ispirati a uno spirito costruttivo e che fanno leva anche sulle competenze dei membri della Commissione in materia di scuola e università. abbiamo ricevuto 117 no. È impossibile che la maggioranza sia stata 117 volte nel giusto e che noi siamo stati 117 volte sbagliati. È statisticamente impossibile e contro la logica; è una testimonianza assoluta di arroganza. Mi dispiace che il ministro Valditara se ne sia andato, ma sicuramente per dottrina di studi saprà perfettamente che l'*hỳbris* è il peccato mortale che porta alla distruzione del politico. Desidero discutere di un aspetto relativamente minore, ma non per questo meno significativo. A proposito dell'avvio dell'anno scolastico, all'articolo 14 si propone di dare la possibilità al personale impiegato all'estero nelle scuole europee, che sono al sesto anno di servizio (quindi in scadenza), di prorogare il rapporto di impiego per altri tre anni. Ricordo che le scuole europee sono state istituite con lo scopo di dare la possibilità ai figli del personale delle ambasciate e dei consolati di continuare il percorso di studi secondo l'ordinamento scolastico originario del Paese di appartenenza. Sono solo 14 queste scuole. scuole. Non voglio entrare nella *ratio* del provvedimento, ma rilevo che gli insegnanti italiani in servizio presso queste scuole sono solo 118. Sì, esattamente 118. E coloro che sono al sesto anno sono 15. Il Senato della Repubblica, signori, sta deliberando su un provvedimento che interessa 15 persone, di cui - forse - solo una o due interessate. mi permetta di dire che non capisco perché non siano stati inclusi i docenti che operano nel sistema di formazione italiana nel mondo, che sono di gran lunga più numerosi (circa 1.000).

in costante aumento; di questi, 3,2 milioni vivono in Europa e nel Regno Unito (Londra da sola conta 375.000 abitanti italiani iscritti all'AIRE, cosa che la pone come ottava città con abitanti italiani, tra Firenze e Bologna). Ebbene, vi parlo per esperienza personale: se un italiano vuol far studiare al proprio figlio l'italiano nel Regno Unito è impossibile; può imparare lo spagnolo, può imparare il tedesco e può imparare il francese, ma l'italiano no.

92 sezioni di italiano nelle scuole internazionali: a questo punto, non ci dobbiamo sorprendere se il 60 per cento degli italiani residenti all'estero non conosce l'italiano perfettamente e non è in grado di interpretare testi e cultura italiani. Si tratta in gran parte di seconde e terze generazioni, giovani che hanno accumulato un patrimonio di competenze e che non torneranno mai più in Italia. Questi giovani non è che non imparano e non conoscono l'italiano per volontà, ma purtroppo per la situazione che si è venuta a creare, cioè per quello che noi abbiamo offerto, che sicuramente è un'ingiustizia. Abbiamo quindi cittadini italiani che non sanno l'italiano e non sanno nulla di cultura italiana, mentre qui abbiamo ragazzi, ragazzi, figli di immigrati nati in Italia, perfettamente integrati, che sanno l'italiano e non sono cittadini italiani. Penso che anche su questo bisognerà riflettere. A questo proposito, sull'avvio dell'anno scolastico per gli italiani all'estero, mi sarei aspettato che qui in Senato, invece di varare un provvedimento che interessa una o due persone, si aprisse un confronto su come potenziare la rete didattica e sul finanziamento degli enti gestori delle scuole parificate, che è insufficiente e arriva sempre in ritardo, mettendone in pericolo la funzionalità e la vitalità. vitalità. Penso che la maggioranza qui, in questa occasione, dimostri ancora una volta che degli italiani che vivono all'estero non le importa assolutamente nulla. Colgo anche qui l'occasione per dire che non ci dimentichiamo che, giusto pochi mesi fa, avete negato a un milione di italiani che vivono in Svizzera e nel Regno Unito di votare alle elezioni europee. Si ignorano i diritti fondamentali di milioni di persone, ma siamo qui ad approvare premurosamente un articolo che interessa al massimo 15 persone. Ora, qui non comprendo di nuovo perché non siano stati approvati gli emendamenti che estendevano gli stessi diritti a tutta la comunità degli insegnanti distaccati nel sistema didattico di formazione all'estero. Presidente, a questo punto mi auguro che questa maggioranza esaurisca presto la lista degli amici e parenti da sistemare e privilegiare e passi a interessarsi e risolvere i problemi dell'Italia e degli italiani.

*(M5S)*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a discutere di un provvedimento pieno di buone intenzioni e di interventi spot, ma svuotato di efficacia, privo di lungimiranza e soprattutto di un progetto a lungo termine per rilanciare il mondo della scuola, dello sport, dell'università e della ricerca. Il provvedimento in esame, approdato quest'oggi frettolosamente dalla Commissione all'Aula, disciplina diverse misure in materia di sport e di lavoro sportivo, nonché la relativa disciplina fiscale, disponendo anche interventi in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di reclutamento del personale docente e infine di università e ricerca, una vera accozzaglia di annunci. In poche parole, il Governo Meloni ha proposto l'ennesimo decreto *omnibus*, in cui si parla di tutto e di niente, pensato male e scritto peggio. Già al principio del 2023 l'Istat, in un *report* sui divari territoriali, così dipingeva lo stato di salute della scuola nel Meridione. nelle scuole del Sud Italia le competenze degli studenti risultano più basse in tutte le discipline e il *gap* aumenta nei diversi gradi di istruzione. Tali fenomeni inediti, se non governati con urgenza, possono far incamminare in Mezzogiorno verso un'involuzione radicale e molto problematica della funzionalità e della sostenibilità della propria struttura sociale. Se non si riesce a porre un freno -concludeva l'Istat nel proprio *report -* le tendenze in atto possono condurre verso un'involuzione progressiva e non sostenibile del capitale umano e di molta parte del Mezzogiorno, che storicamente è stato il suo principale patrimonio. Qual è stata la risposta del Governo? Tentare di introdurre le gabbie salariali nel mondo della scuola, come riferito e auspicato dal ministro Valditara, che arrivò a ipotizzare l'ingresso di soggetti privati per sostenere economicamente gli stipendi differenziati dei docenti settentrionali. Ebbene appare evidente che il ministro Valditara è più interessato a favorire taluni interessi privatistici invece che a restituire al nostro sistema scolastico il ruolo di presidio sociale ed educativo. Infatti avrebbe potuto implementare la scuola a tempo pieno e aggiungere nuove discipline educative e formative, quali il teatro o la cinematografia. Ebbene il forte dimensionamento scolastico, registratosi soprattutto in molte Regioni meridionali, ha di fatto creato mega istituti nei quali risulta particolarmente difficile mantenere un adeguato rapporto scuola-famiglia, elemento fondamentale per la lotta alla dispersione scolastica e alla criminalità minorile. Pensate che in Sardegna l'accorpamento è arrivato a coinvolgere fino a 40 Comuni con una unica dirigenza, cancellando posti di lavoro fra personale ATA (assistente tecnico amministrativo) e docenti in materia definitiva. Presidente, onorevoli colleghi, certamente non potrò soffermarmi sull'intero articolato, però intendo accendere un faro su talune criticità che non possiamo sottacere. Per cominciare, i tempi dettati dalla conversione in legge sono stati così esigui che questa maggioranza non è riuscita ad ascoltare attentamente tutte le categorie interessate, incassando tuttavia diverse bocciature che non sono state prese minimamente in considerazione. Cisl scuola - conferire a soggetti esterni alla scuola, a prescindere dalla loro competenza e senza alcuna garanzia di obiettività, il potere di esprimere una valutazione con dirette ricadute sul lavoro di chi insegna. Mi riferisco in particolare alle misure riguardanti la possibile conferma di supplenti sul posto di sostegno anche in base al gradimento espresso dai familiari dell'alunno seguito. Mi chiedo quali competenze possa avere un genitore che ha una sola preoccupazione - la presenza - senza considerare i contenuti dell'azione educativa e la sua efficacia. Si annulla così la qualità dell'insegnamento e si trasformano le ore di lezione in un vero intrattenimento da salotto, ma soprattutto la scelta viene affidata a criteri soggettivi e clientelari, annullando del tutto una valutazione scientifica tecnica, quindi oggettiva. Non solo, in questo modo si consegna alle famiglie un potere che va ben oltre il diritto di esigere per i propri figli la migliore qualità del servizio. La norma ignora evidentemente che l'insegnante di sostegno non agisce isolatamente, bensì in un rapporto di interazione con l'intero *team* docente. Non è pertanto con queste modalità che si garantisce la continuità didattica, minata in realtà alla radice dalla troppo estesa precarietà del lavoro. Come poi evidenziato nella questione pregiudiziale, si prefigura in tal modo una sorta di chiamata diretta dei docenti di sostegno in contrasto con l'articolo 3 e i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 97 della Costituzione, nonché in palese violazione delle procedure di reclutamento e conferimento delle supplenze. Ebbene, su questa materia, come parimenti su ciò che attiene ai nuovi percorsi per il conseguimento del titolo di specializzazione, servono interventi strutturali, non misure *spot* o dettate dall'emergenza affinché non emergano iniquità o disparità di trattamento. Altra menzione di criticità meriterebbe l'articolo 6, laddove si conferisce la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno, non solo in via ordinaria, tramite i percorsi di tirocinio formativo attivo erogati dalle università, ma anche in via straordinaria, tramite percorsi da trenta crediti formativi universitari erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Non solo, ma è un vero e proprio regalo a chi non ha le competenze e riconosce di fatto un ruolo non rispondente alle competenze. Al netto di un chiaro *assist* al mondo privatistico, è evidente che questo provvedimento finirà per generare un *vulnus,* evidenziando una spaccatura tra coloro che frequenteranno il nuovo percorso per i trenta CFU, con minore durata e impegno solo *on line*, e il lavoratore, già iscritto al nono ciclo dei TFA universitari, che rientrano nella riserva del 35 per cento, di durata di nove mesi e che fanno fronte a una quota di iscrizione per un percorso da sessanta CFU in presenza. Genera perplessità anche l'introduzione del docente per stranieri nelle classi con un numero di alunni stranieri pari o superiore al 20 per cento. Se l'obiettivo è garantire, attraverso la conoscenza della lingua italiana, una reale eguaglianza tra tutti gli studenti, nei fatti si genererà l'effetto opposto, attraverso una ghettizzazione tra i ceppi di studenti, alimentata da un corpo docente separato che farà percepire lo straniero come un'entità a parte. Tutto ciò a tacere dell'articolo 15, che istituisce l'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, termine già più volte oggetto di proroga a partire dal 2022, e che assume le fattezze di un ingiustificabile perenne rinvio di una disposizione da cui dipende la vita di migliaia di ricercatori italiani. Sono sincera, ci aspettavamo l'approvazione di emendamenti correttivi, sia in fase di prima lettura alla Camera sia in Senato. Il decreto-legge è rimasto pressoché identico nella sostanza, a fronte di una totale indifferenza dell'Esecutivo rispetto alla possibilità di migliorare un testo che rema in direzione ostinata e contraria rispetto ai reali interessi degli studenti e dei docenti, degli atleti e dei disabili. Si registra solo una piccola modifica rispetto al punteggio minimo necessario per superare sia la prova scritta sia quella orale del prossimo concorso docenti, cosicché un emendamento che è stato approvato solo in parte ha rivisto la classe di concorso e posizione.

Bisogna prendere atto che sono le scuole i luoghi in cui si formano le nostre coscienze, non solo sul piano accademico, ma anche in quello sociale e culturale. È nella scuola che nasce un senso di appartenenza e l'amore per il proprio Paese, e si coltivano i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile. Però, se la scuola, così come le università, diviene luogo di repressione del dissenso e di mancanza di dialogo e confronto, allora stiamo fallendo nel nostro compito di formare cittadini consapevoli e responsabili.

il testo oggi in discussione in quest'Aula, uscito dal voto di fiducia alla Camera dei deputati, che ha azzerato ogni confronto, è quello è che ormai potremmo definire l'eterno ritorno ai decreti *omnibus*. Con quello di oggi siamo al decreto numero settantasette. In un anno e mezzo di legislatura è un *record* negativo che non si era mai visto nella storia repubblicana, quello dell'abuso del potere esecutivo su quello legislativo del Parlamento.

che tratta argomenti riconducibili a ben quattro Ministeri diversi: dallo sport al sostegno scolastico fino all'università. Un insieme di norme e modifiche che costituiscono un mosaico in cui mancano sempre tasselli per un quadro organico. Presidente, è il caso di questo decreto-legge, ed entro così nello specifico del provvedimento, concentrandomi su alcuni aspetti a nostro parere di particolare criticità, a partire dalle modifiche che vengono introdotte per gli insegnanti di sostegno. In questo caso, il Governo sembra individuare il problema che potremmo riassumere nella necessità di incrementare il numero di docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, ma sbaglia completamente le soluzioni. I numeri degli insegnanti di sostegno, la carenza e l'alto tasso di precarietà sono stati spiegati in audizione da diversi auditi, ma in particolare dalla CGIL. Nell'anno scolastico 2023-2024 si è arrivati a quota 103.000 insegnanti a tempo determinato e oltre 13.000 posti sono rimasti scoperti. Davanti a questi numeri, ci si sarebbe aspettati una programmazione seria a partire dal fabbisogno regionale, valorizzando l'esperienza formativa del tirocinio formativo attivo per il sostegno. Niente di tutto questo. Davanti al problema ci si inventa una nuova strada, che rischia di generare ancora maggiore confusione, affidando il percorso di specializzazione di docenti di sostegno e riducendo la formazione a 30 crediti formativi universitari (CFU). Diversi canali di reclutamento rischiano di creare insegnanti di serie A e di serie B, incidendo sulla qualità della formazione e della conoscenza. A proposito di INDIRE, questo pacchetto di norme fa anche peggio, perché avvia a tutti gli effetti il commissariamento dell'Istituto, facendo decadere tutti i suoi organi e istituendo un commissario. È la plastica rappresentazione della volontà di questo Governo di considerare gli enti di ricerca come strumenti per le proprie esigenze, di voler prendere il controllo diretto sulle filiere della conoscenza. Sul sostegno, voglio sottolineare le modifiche contenute all'articolo 8 di questo provvedimento, che mirano a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posti di sostegno tramite la conferma, su richiesta delle famiglie. per come sono state scritte, rischiano invece di cristallizzare la precarietà lavorativa e di essere l'avvio dello smantellamento del sistema di reclutamento basato sulle graduatorie, sulla trasparenza e sulle regole certe, sostituendolo con un meccanismo che metta al centro una sorta di chiamata diretta da parte della dirigenza e delle famiglie. In Commissione abbiamo cercato, con alcuni emendamenti, di dare una soluzione a questo problema garantendo sicuramente la continuità per gli alunni disabili. Purtroppo - lo dico con amarezza - non stupisce che il Governo non abbia messo in campo nessuna delle soluzioni strutturali richieste, preferendo piuttosto scorciatoie e soluzioni temporanee che creano solo ingiustizie e disparità. non stupisce perché stiamo assistendo sin dall'inizio della legislatura a questo modo di fare su tutti i temi. Durante il confronto in Commissione, abbiamo chiesto una proposta seria e sostenibile, che sia centrata sul modello di inclusione della scuola italiana e che sappia partire dalla partire dalla necessità e dall'urgenza di stabilizzare i docenti di sostegno, riconoscendone il ruolo fondamentale che hanno per l'educazione degli alunni con disabilità. Il nostro sistema scolastico ha un insieme di strumenti e pratiche che garantiscono l'inclusione di tutte le alunne e gli alunni delle scuole italiane, frutto di un sistema complesso che richiede l'attenzione del legislatore per assicurare il miglior funzionamento. Con queste norme si sbaglia la strada e si mette a rischio un pezzo importante del sistema scuola. Se pensiamo a queste modifiche accanto alla legge sull'autonomia differenziata, che avete già approvato, il rischio concreto di arrivare ad uno smantellamento del sistema di istruzione è tragicamente alle porte. Norme parziali, signora Presidente, che producono diseguaglianze e aumentano i problemi invece di risolverli. Anche sulla importante questione dell'integrazione degli studenti con *background* migratorio siete stati capaci di approvare una legge a metà: l'accoglimento alla Camera dell'emendamento proposto dall'ANCI che ampliava le categorie di studenti che possono ricorrere al supporto del docente di italiano per stranieri sembrava essere il segnale di un percorso giusto, ma in realtà la misura che oggi arriva in Senato è ancora fortemente incompleta, perché manca di un sistema di certificazione linguistica uniforme a livello nazionale, perché quell'organico di potenziamento con docenti di lingua italiana per stranieri dovrebbe essere non una misura provvisoria, ma un caposaldo per ogni politica di inclusione. Questo è un punto decisivo, perché questa norma arriva a poche settimane di distanza dall'uscita infelice del ministro Valditara sulle classi separate per stranieri: una follia, perché quelli che voi chiamate stranieri sono ragazze e ragazzi nati e cresciuti in Italia, che non hanno la cittadinanza perché manca ancora una legge che consenta di riconoscerla. L'idea di integrazione limitata all'apprendimento della lingua italiana attraverso momenti separati è riduttiva e controproducente, presenta profili di discriminazione e soprattutto, come già visto in altri esempi in passato, non funzionerà. Presidente, in questi pochi minuti di intervento è spesso tornata la parola «inclusione», perché è attorno a questo principio che prende forma il modello della scuola italiana; un sistema che, pur nelle difficoltà e nella necessità di costante aggiornamento, rappresenta un caposaldo del nostro Paese. Le norme confuse del decreto-legge in esame, accanto ai propositi e alle dichiarazioni arrivate nei mesi da parte degli esponenti del Governo Meloni, sembrano andare nella direzione opposta, per costruire un modello sbagliato e punitivo (penso alla pessima norma sul voto in condotta che ci avete presentato), divisivo e a svantaggio degli insegnanti. La scuola è l'immagine di una società, il luogo nel quale inclusione e dialogo sono pilastri dello stare insieme; voi volete distruggere questo modello, ormai è chiaro. Noi continueremo a batterci contro il vostro modello: non c'è nulla che sia più ingiusto quanto il fare parti uguali fra disuguali, come diceva don Milani. sfida, la vostra ossessione sembra essere quella di fare leggi per pochi che danneggiano molti e questo incide su una società che si costruisce sempre più su diseguaglianze di sapere, di conoscenze e di opportunità per tutte e tutti.

intanto vorrei dire ai colleghi che la decretazione d'urgenza, ovviamente, rappresenta l'*extrema ratio* per i provvedimenti che il Governo ritiene urgenti, come è testimoniato dai contenuti. su questo vorrei intrattenermi, perché è evidente che i toni in Aula siano legittimamente diversi da quelli che abbiamo in Commissione, ci mancherebbe: toni differenti, anche ingiusti, apocalittici, strumentali, ma in Aula si sa che i toni sono questi.

dire - che abbiamo trovato tante urgenze da risolvere, quindi se il Governo ci mette mano in fretta, senza aspettare i tempi ormai lunghi delle ordinarie procedure parlamentari, è un bene per il Paese.

che gli interventi che si realizzano sono due pezzi di un mosaico, di una riforma complessiva che stiamo man mano individuando. Forse la riforma ancora la stiamo individuando perché stiamo ancora finendo di ascoltare tutti i personaggi che fanno parte del mondo del calcio e che ci lavorano.

lui stesso a chiudere, se noi vorremo, in Commissione, tutto il nostro lavoro di audizioni, ma che sarà ben felice di raccogliere quello che sarà un atto di indirizzo o ciò che decideremo di fare, per poterlo poi adottare a livello governativo. Quindi mi sento rafforzato, perché quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato già accolto nel primo provvedimento utile sullo sport nello *slot* che era disponibile per realizzare un governo sullo sport.

la riforma del calcio, che noi abbiamo affrontato già da diversi mesi, non viene aggravata dal pessimo risultato dei recenti europei, ma nasce da lontano: se n'è già parlato, soprattutto ne hanno parlato le componenti del calcio, senza avere però la capacità di autoriformarsi. autoriformarsi. Quindi gli anni passano, ma i risultati non arrivano. Si tratta di un settore non solo sportivo: si dice che è un'industria di emozioni collettive che che genera partecipazione e passione, ma, per noi che ci occupiamo di politica e di trovare delle misure adeguate, bisogna sempre ricordare, per non svilire l'argomento, che è un settore che produce un indotto di 11 miliardi

L'urgenza è stata anche accelerata, perché recentemente, come abbiamo capito, la volontà di rinnovare le cariche della presidenza del consiglio federale della FIGC con le attuali norme non avrebbe dato la possibilità di intervenire neanche alla Commissione con una riforma, se non successivamente.

anche per fare in modo che ospitino oltre ai tifosi anche le famiglie o iniziative ludiche e culturali per tutta la settimana. Insomma, occorre ripensare il calcio in modo che si concepisca non solo come una somma di associazioni sportive, ma anche come un *asset* industriale importante per questo Paese.

rispetta il pareggio di bilancio. Non a caso, in questo provvedimento c'è un articolo che riguarda la maggiore trasparenza degli organismi di controllo. in esame si inserisce nel nostro lavoro per una valorizzazione del calcio italiano nel suo complesso, come fatto anni fa dalla Premier League inglese, che ha saputo fare sistema. Per dare credibilità a questo sistema dove girano tantissimi interessi e investimenti, per il Governo era necessario - e io condivido inserire la norma che individua un'autorità indipendente composta da profili di altissima professionalità. Si sottolinea strumentalmente che saranno nominati dal Governo, ma si omette che saranno composti da profili di altissima professionalità. dovrà certificare finalmente la regolarità economica e finanziaria delle società di calcio. Noi faremo il nostro lavoro in Commissione e sappiamo che e sappiamo che sarà accolto dal Ministro dello sport e da tutto il Governo. Lo abbiamo fatto del resto all'unanimità in Commissione più volte sul tema dello sport per l'articolo 33, ma anche sui Giochi della gioventù, che speriamo l'altro ramo del Parlamento porti a compimento.

Evidenziando l'importanza di una visione complessiva del sistema, abbiamo inserito - questo è un altro punto fondamentale che ha suscitato molte polemiche, come sentivo dai colleghi del MoVimento 5 Stelle - le norme sull'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato dal sistema sportivo della Lega di Serie A. Ricordo ai colleghi che nessuno ha chiesto alla Federazione una percentuale di maggioranza e di minoranza, ma solo un indirizzo di allargamento delle rappresentanze della Lega di Serie A, sul quale si basa tutto il principio di mutualità, che nessuno ha sottolineato. Voglio ricordare che le nostre regole, che sono datate, si basavano su un ordinamento sportivo composto da associazioni sportive. Adesso si parla di società quotate in borsa, una decina delle quali, in Serie A, sono proprietà di finanziarie internazionali; si tratta di un mondo completamente nuovo rispetto a quello che abbiamo normato ben vent'anni fa. Quindi un adeguamento è necessario.

Ci saranno pesi e contrappesi, che dovranno scegliere direttamente gli addetti ai lavori all'interno delle loro federazioni.

il popolo italiano aveva già scelto un'altra maggioranza e ancora si doveva praticamente firmare questa riforma. A onor del vero il ministro Abodi, avendo dato la sua parola,

la nomina del commissario straordinario di Milano Cortina 2026, per la realizzazione di talune opere, e il riconoscimento finalmente, dopo diciassette anni, della NADO (il nostro istituto antidoping), che ci invidiano anche altri Paesi. Grazie Onorevoli senatori, voglio replicare ad alcuni punti che mi paiono, nella loro *vis polemica*, non corrispondenti alla realtà degli emendamenti approvati e del testo presentato dal Governo. E, soprattutto, non sono rispondenti agli effetti degli emendamenti approvati e del testo presentato dal Governo. Iniziamo con l'emendamento parlamentare relativo ai dirigenti scolastici. Non è vero che vi sarà uno scavalcamento da parte dei vincitori del concorso riservato a danno dei futuri vincitori del concorso ordinario, semplicemente perché il concorso ordinario non si è ancora concluso. Quindi, i vincitori del concorso ordinario potranno prendere servizio soltanto dal prossimo anno scolastico. Dunque, abbiamo programmato che ci saranno i posti necessari per dare copertura al concorso ordinario che si sta svolgendo. si sta svolgendo. L'alternativa sarebbe stata quella di affidare a dirigenti reggenti, e cioè estendere l'istituto della reggenza che proprio voi avete più volte criticato in passato e che non garantisce la qualità

questo provvedimento, che non toglie alcun diritto e alcuna prerogativa a coloro che si sono iscritti al concorso ordinario. C'è poi il problema della specializzazione dei docenti precari sul sostegno. lo dico con grande pacatezza - che a voi non sfugga la realtà e mi fa piacere che, pur polemizzando, la senatrice Malpezzi in qualche modo abbia riconosciuto la gravità del problema. Vi do soltanto un dato che credo sia testimonianza di una situazione drammatica: al Nord 10.897 posti 13.133 non saranno assegnabili per carenza assoluta di candidati specializzati. Sappiamo che ci sono 85.000 docenti precari sul sostegno che non hanno la specializzazione e che il sistema universitario non può e non è in grado di formare. Dunque, l'alternativa è che ai nostri ragazzi con disabilità

di almeno 30 crediti formativi. Qualcuno ha detto che sarebbe stato inferiore ai 30 crediti e da qualche parte ho addirittura letto 10 crediti. È falso, mai detto questo. La legge specifica almeno 30 crediti formativi. Per la definizione di questi 30 crediti sarà coinvolto direttamente l'Osservatorio per l'inclusione, così come non accade per il TFA. il TFA. Anche da questo punto di vista, credo che, se non fossimo intervenuti, non avremmo dato l'opportunità ai nostri ragazzi di avere docenti sempre più preparati e specializzati. D'altro canto, è stata criticata anche la norma che coinvolge le famiglie e che consente loro di chiedere la continuità didattica. Si tratta di una norma che le associazioni

bonaria e veramente benevola terminologia - anzi, cari onorevoli, conosciamo l'articolo 30 della Costituzione, che attribuisce ai genitori il diritto-dovere di istruire, educare e formare i propri figli? E allora i genitori non sono i privati che entrano nella scuola. Se la scuola - come io sostengo, come noi sosteniamo e come questo Governo sostiene - deve avere al centro innanzi tutto la persona - perché è questo che la Costituzione vuole

Semmai, la necessità di un'accelerazione è dovuta anche a una sentenza del Consiglio di Stato, per risolvere un problema che oggettivamente si trascinava

che riguarda migliaia e migliaia di precari che insegnano nella nostra scuola. Da questo punto di vista, allora, non dobbiamo dimenticarci che ci sono una giurisprudenza europea, norme europee e una giurisprudenza italiana, che ci obbliga

di abilitarsi con il raggiungimento di un numero importante di crediti - tenendo conto oggettivamente che all'estero non vi è un sistema simile a quello italiano e, quindi, è necessario

per cento dei ragazzi stranieri di prima generazione abbandona la scuola perché non ha le competenze necessarie e ha difficoltà a proseguire, per carenze innanzi tutto nella conoscenza della lingua italiana.

poi, già dal prossimo anno scolastico, con una formazione obbligatoria pomeridiana per quei ragazzi che non conoscono adeguatamente la lingua italiana o che non la conoscono affatto; infine, con la formazione e il reclutamento di appositi insegnanti specializzati per insegnare l'italiano agli stranieri. Questa è una misura di grande inclusione. Ragazzi, cari onorevoli, se un giovane non conosce la lingua italiana, non può neanche integrarsi, non può conoscere la cultura italiana;

un abbandono così elevato fra gli studenti stranieri di prima generazione. Credo allora che forse un intervento di questo tipo avrebbe dovuto essere accolto con maggiore condivisione da parte di chi ha veramente a cuore il problema della integrazione dei giovani stranieri nel nostro sistema e nella nostra società. Concludo con una smentita drastica nei confronti della senatrice che è intervenuta precedentemente affermando che io avrei dichiarato o auspicato che i docenti del Nord vengano pagati dai privati. Questa affermazione è totalmente falsa. Non ho mai dichiarato qualcosa di simile: ho semplicemente auspicato che anche i privati, come accade in tutto il mondo, facciano la loro parte, contribuendo a finanziare la scuola italiana. La quota

privati, agli imprenditori, a coloro che hanno le disponibilità finanziarie e l'interesse economico per far sì che la nostra scuola possa essere sempre più dotata di risorse, sia risorse, sia opportuno e necessario, fermo restando che il Governo sta facendo la sua parte come ha dimostrato con i due contratti, di cui il primo è già siglato e il secondo abbiamo in animo di siglare entro quest'anno. Tali contratti certamente contengono risorse mai prima d'ora destinate agli aumenti degli stipendi del personale della scuola, mai prima d'ora realizzate. Grazie per l'attenzione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. Grazie finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. Commissione identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

però devo confessarle che è irrituale anche questa fiducia. Siamo alla sessantesima fiducia su 72 decreti legge. È irrituale perché è una fiducia sulla maggioranza. Le opposizioni Le opposizioni avevano dato la disponibilità alla maggioranza di entrare nel merito di alcune questioni, ovviamente

relatore Marcheschi, lei giustamente ha rivendicato l'idea originaria. pochi secondi solo per far notare ai miei colleghi Presidenti dei Gruppi di maggioranza che cosa stiamo facendo. Il relatore Marcheschi ci ha presentato un provvedimento sullo sport.

per evitare che i Gruppi di maggioranza si esprimano. Questo è il tema: è stata posta una questione di fiducia sulle posizioni di Forza Italia che divergono da quelle degli altri partiti di maggioranza.

tre disegni di legge di conversione dei decreti-legge, due dei quali sono ancora in alto mare e non arriveranno qui in Aula fino a giovedì o venerdì. Quindi, da adesso fino a giovedì mattina non capisco perché non vi sia il tempo per votare i 160 emendamenti

sottolineando lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Io so che anche in passato si è molto utilizzata la decretazione d'urgenza e il voto di fiducia, ma stiamo raggiungendo livelli veramente mai visti prima. Sappiamo anche che i decreti da

Noi stiamo assistendo a continui voti di fiducia e a giorni di non lavoro dal punto di vista parlamentare, perché sui decreti che ingolfano la discussione non ci sono mai i pareri e alla fine si si pone la fiducia. Questa è la dimostrazione di qualcosa che non funziona. Io sono d'accordo con quello che diceva il presidente Boccia,

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in materia di sport, alunni con disabilità e avvio dell'anno scolastico nel testo approvato alla Camera dei deputati. La seduta riprenderà alle ore 16,30 con le dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. In apertura della seduta di domani si terrà un dibattito sulle prossime elezioni in Venezuela, i Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Si proseguirà con la discussione del decreto-legge in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Qualora il Governo ponesse la questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di attribuire complessivamente 55 minuti per la discussione sulla fiducia in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama. Sospendo la seduta.

contiene alcune misure estremamente importanti che obiettivamente, a mio personale avviso ma non solo mio, meritavano di essere approfondite e soprattutto condivise con provvedimenti singoli e dedicati. Invece le forze politiche non sono state coinvolte adeguatamente come ci saremmo aspettati e ci troviamo di fronte di nuovo a una questione di fiducia posta dal Governo che impedisce di fatto un sano confronto. Questo provvedimento arriva tecnicamente blindato dalla Camera, imponendo quindi anche al Senato, a tutti noi, semplicemente di ratificare quanto si è già deciso nell'altro ramo del Parlamento.

evidenziando le numerose criticità contenute in questo provvedimento, ma è superfluo dire che sono stati respinti. Il decreto-legge in esame parla di sport, scuola e disabilità, tutti temi di notevole rilevanza che meritavano però un lavoro puntuale puntuale e molto più condiviso. Il tempo a mia disposizione mi impone di correre ma, per quanto io ami la corsa, in questo caso specifico avrei preferito andare molto più lentamente per approfondire meglio i temi. Proverò quindi ad essere sintetica ricordando alcuni punti chiave presenti in questo testo e analizzando brevemente anche le principali finalità che esso vuole disciplinare, peraltro peraltro coinvolgendo anche più di tre o quattro Ministeri. Il primo è lo sport, con due articoli dedicati al funzionamento degli organismi sportivi e una commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Al di là delle polemiche di questi giorni, guardiamo con obiettività la questione. Di fatto, si istituisce un altro organo di controllo e, pur se volessi comprenderne le buone ragioni, non posso non manifestare perplessità sul rischio di ledere quel principio di autonomia previsto dall'ordinamento sportivo e anche ribadito dalla Corte costituzionale. Con questo provvedimento di fatto si dà vita a un'altra forma di controllo statale su società di capitali private. scelta opinabile, ma direi che non vedo i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustifichino l'emanazione di un decreto-legge. C'è poi la parte che rivede le regole relative all'elezione degli organismi sportivi per l'intervento emendativo sull'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999. Può anche essere giusto e condivisibile eliminare la previsione del *quorum* rafforzato di due terzi dei voti validamente espressi dai consiglieri federali e i consiglieri regionali. Quello che non si capisce è perché queste stesse regole oggi previste per gli organismi sportivi, compresa la parte legata al limite dei mandati, non valgano anche per gli organi territoriali e periferici di enti come il CONI, nonché il CIP. Sono discriminazioni che non trovano nessuna giustificazione giuridica né politica. Occorre secondo me anche ricordare - vale la pena farlo proprio in quest'Aula - che i componenti degli organi territoriali del CONI e del CIP vengono eletti e operano a titolo gratuito e volontario; sono spesso difficili da sostituire, esattamente come i componenti degli organi federali territoriali. Sarebbe stato saggio e opportuno a questo punto prendere in considerazione una volta per tutte la possibilità di uniformare, così come è avvenuto per le federazioni, anche la durata e le nomine di tutti gli organi del CONI e del CIP dai vertici ai territori, come prevedeva l'emendamento, e stabilendo anche per loro la rielezione a fronte dei due terzi, del 66 per cento non esiste una necessità giuridica di uniformare le situazioni, ma ci sarebbero molte buone ragioni di opportunità per fare quello che chiedevo. La mia proposta è un giusto compromesso tra continuità e rappresentatività, con la fisiologica alternanza della democrazia. Anche questa è stata un'occasione persa. Un punto ulteriore di estrema importanza presente nel decreto è la regolamentazione degli insegnanti di sostegno. Come è noto - lo abbiamo già detto anche in discussione generale - i dati dell'Istat ci dicono che ogni anno sono in aumento i bambini con disabilità: per cento in più rispetto all'anno precedente. Un aumento, purtroppo, che non è al passo con il sistema della formazione dei docenti di sostegno, in quanto le università italiane non sono ancora pronte per offrire una risposta adeguata. È per questo che il Ministero, con questo provvedimento, decide di aggiungere INDIRE alle università, come ulteriore canale di formazione per garantire continuità didattica. Questo ci può anche stare, però il meccanismo adottato non è del tutto idoneo a raggiungere lo scopo e ci dispiace che anche in questo caso le nostre proposte, che erano volte a semplificare le procedure, non siano state ascoltate. Avevamo chiesto di prevedere il libero accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno a chiunque possegga un titolo di studio coerente con la classe di concorso e ancora di prevedere, per coloro che sono in possesso di un titolo estero e che al contempo hanno frequentato con successo un corso TFA sostegno presso atenei italiani, con enormi sacrifici personali ed economici, di sostituire i corsi attivati dall'INDIRE, previsti dall'articolo 7 di questo decreto, poiché hanno certamente acquisito una specializzazione completa, al pari dei docenti. Questo gli avrebbe consentito consentito sicuramente di superare le possibili mancanze del corrispondente titolo estero. Infine, c'è il tema importante relativo all'avvio del nuovo anno scolastico, quello della residenza degli studenti. Come Azione, avevamo proposto di incaricare il commissario straordinario previsto nel decreto per attivare e individuare iniziative volte a garantire la ristrutturazione di edifici pubblici e privati in tempi brevi, anziché impegnare i fondi solo per la costruzione di nuovi edifici. Tutte proposte semplici e di buonsenso, che certamente, se fossero state maggiormente condivise, avrebbero rappresentato un grande e importante gol per l'intero Parlamento. Alla luce di quanto ho appena esposto sinteticamente (ci ho provato) e avendo scelto di porre la questione di fiducia, noi non possiamo che esprimere un voto contrario, auspicando che in futuro si possa trovare più rispetto per la funzione che questa Assemblea è chiamata a svolgere. Presidente, prima di concludere, mi permetta di rilanciare da quest'Aula il mio personale grandissimo in bocca al lupo a tutta la nazionale olimpica e paralimpica, che è partita o che sta per partire per gli imminenti giochi di Parigi.

Io non so dove ha sede la memoria in questo complicatissimo strumento che è il cervello, che ho cercato di studiare, ma penso di conoscerne un miliardesimo. So però che, quando sento parlare di sport e di disabilità, penso a me - scusate il narcisismo - perché ero bravo. Ho imparato, prima ancora che a camminare, a nuotare nelle dolci spiagge e acque di San Benedetto del Tronto. Poi ho cominciato a camminare in qualche modo un po' storto; qualche volta il segno della corsa erano lividi e croste sulle ginocchia, segno di libertà. Ho cominciato a fare sport e anche a vincere: questa bellissima sensazione di fregare, a pallavolo o a pallanuoto, a ruzzica o a rubabandiera, i cosiddetti normali. Porca miseria, che meraviglia! Però, c'è sempre un però. Quanto ho sofferto rimanendo a casa, perché a scuola ho potuto fare solo alcuni anni del liceo, ma anche allora esonerato dallo sport. Beh, lì mi sono sentito veramente, forse per la prima e l'ultima volta, disabile.

si viene offesi, soprattutto per chi lo dice, sentendosi nominare come fascisti. Ma forse lo dice lo dice chi lo è, perché nego che una persona che ha sempre combattuto contro le leggi razziali e contro tutto quello che negava, prima ancora che gli altri (un po' di egoismo *ce vo'*, quando *ce me stesso, è segno proprio di ignoranza psicoaffettiva, prima ancora che politica, una mancanza di rispetto. Quando si manca di rispetto non si fa politica, ma ci si mette dalla parte della colpa, non del torto. Detto questo, credo che parlare di sport, disabilità e allargamento delle possibilità di sostegno sia cosa buona e giusta. Ieri,

senza specializzazione. Insisto: gli insegnanti di sostegno non sono solo per la persona con disabilità,

quindi riguarda tutti. Dove esiste un buon insegnante di sostegno, anche con un bambino con gravi problematiche di disabilità, tutti stanno meglio, perché c'è un'educazione alla diversità e all'accettare l'altro accettando se stessi, che forse oggi è il compito più difficile che abbiamo di fronte, anche in quest'Aula. Ben venga allora questo provvedimento, non solo per quello che prevede, ma anche per quello che dice e fa discutere: facciamolo con serenità; facciamolo per chi non ha voce in capitolo oggi, perché è fuori da quest'Aula ed è fuori persino dalla scuola per mancanza di sostegno, per mancanza di cultura e per mancanza del darsi generosamente all'altro, sentendosi non inferiore, ma normale nell'accettare la propria diversità e quella degli altri (e forse qua dentro ci vorrebbe un sostegno per qualcuno, che vede l'altro non come avversario - che va sempre, sempre, sempre rispettato - ma come nemico da distruggere con l'arma più potente che abbiamo, che non è la bomba atomica

Poi, con l'ottimo ministro Abodi spero che ci sia una conoscenza che diventi amicizia. Vorrei concludere questo intervento un po' sconclusionato per l'emozione, ma anche per l'età, dato che ci azzecco sempre meno (anche se, vedete, proprio nell'età avanzata la memoria cresce: qualcuno dice che è un simbolo di patologia, io dico che è un dono ricordare meglio le cose belle e anche le brutte, in questo clima così complicato, perché il buono vince sempre).

Siamo conoscenti affettuosi da una vita; quando io ero al sindacato, lui aveva sotto la sede una esposizione di auto meravigliose. È sempre stato legato al bello, al bello rispettoso. Mi ha detto: Antonio, se posso permettermi, ricorda, proprio oggi che sono alla presidenza del CONI, che quando si parla di sport e disabilità, si parla anche di pace. In questo periodo, dove si parla tanto di questi simboli

parlare di sport e disabilità è parlare di pace, di una sfida meravigliosa, dove non esistono vinti e vincitori, esiste un progresso determinato dalla bontà, dall'accettazione dell'altro, ma anche un sostegno tecnico al sistema, soprattutto nelle gare, nelle paralimpiadi e nelle olimpiadi, in classe, dove si esercitano ogni giorno le olimpiadi più importanti della nostra vita. Ecco, io sono commosso, nel senso che mi muove un'emozione enorme nominare disabilità e normalità, nel senso più dolce del termine, scuola e sport. È davvero una sfida meravigliosa che dovrebbe farci sentire oggi orgogliosi di discutere questo argomento. Ringrazio il Presidente, i membri del Governo, i colleghi e il relatore.

anch'io mi associo prima di tutto agli auguri, rivolgendo un in bocca al lupo ai nostri italiani che inizieranno questa bellissima avventura

ben sottolineato da alcuni interventi, è un decreto *omnibus* che mette assieme tanti temi di rilevanza di complessità che avevano bisogno di essere necessariamente elaborati in modo diverso. Per quanto riguarda lo sport *in primis*,

Avevamo la necessità di affrontare una riforma organica dello sport, come abbiamo detto anche in altri momenti del dibattito parlamentare. Lo sport infatti soltanto il calcio, che pure sicuramente è una parte importantissima di una riforma necessaria.

che significa davvero ricerca di nuovi talenti importanti tra i nuovi italiani. Ci lamentiamo sempre di non avere vivai, ma questo *ius soli* sportivo non lo vogliamo poi portare avanti nelle Aule parlamentari e nel Governo. Certamente c'era la necessità, ma non attraverso un emendamento, di affrontare anche il giusto tema di come si arriva alle votazioni all'interno degli organismi dirigenti delle federazioni sportive. Ma anche questo tema è affrontato così, attraverso un emendamento di maggioranza, senza un confronto dialettico necessario, che ci sarebbe stato, con tutti vi è il grande tema di che cosa vogliamo fare, tra professionismo e dilettantismo, rispetto al mondo del volontariato nello sport, di come affrontare lo sport all'interno delle scuole. di un tema importantissimo: l'attività, il movimento, lo sport come prevenzione e come farmaco anche nel contrasto di tante malattie croniche, a cominciare dai bambini più piccoli. Questi sono i temi che noi avremmo voluto vedere, non all'interno di un decreto *omnibus*, ma in una riforma organica dello sport, che significa anche cultura sportiva, che significa impianti sportivi non fatiscenti come quelli che abbiamo, anche perché abbiamo

come affrontiamo il tema di genere all'interno delle società e delle federazioni sportive, basandosi sempre sul merito, sui talenti che noi abbiamo. Questi sarebbero stati i temi che avremmo voluto affrontare con voi, anche in termini di lavoro sportivo, di posti di lavoro e anche di nuove professioni all'interno dello sport. Abbiamo molti disegni di legge che potevano essere tranquillamente affrontati sia dal Parlamento che in un confronto con il Governo. Poi c'è il grande tema

che vede delle misure su cui possiamo anche essere d'accordo, ma che sono misure tampone. Anche qui c'era, invece, la necessità di avere una riforma organica per quanto riguarda l'inclusione scolastica per gli alunni disabili. Questo significa, per esempio, più formazione e più insegnanti di sostegno, a cominciare dalle classi dei più piccoli; un ascolto e un dialogo permanente tra docenti e famiglie. Spesso le due istanze non si incontrano, perché c'è la necessità di andare a lavorare, di rinnovare anche il mondo della scuola attraverso un coinvolgimento maggiore sia degli alunni che delle famiglie. Anche questo punto, purtroppo, ancora una volta è stato toccato in maniera emergenziale, quando invece c'era la necessità di mettere mano ad un lavoro costante, permanente, anche con delle risorse adeguate, mettendo assieme e lavorando anche sul potenziamento dei privati. Penso anche al tema delle scuole paritarie e a tanti temi che potevano essere affrontati in una riforma organica, fino ad arrivare al tema

A noi dispiace, perché dobbiamo fare, così come è stato fatto egregiamente dai colleghi del Gruppo di Italia Viva anche alla Camera, Camera, una considerazione di metodo. Ancora una volta vogliamo mettere in evidenza l'umiliazione del Parlamento e della democrazia parlamentare. Questa è la sede in cui si approfondiscono e si discutono i disegni di legge e nella quale si può trovare anche una trasversalità su molte questioni. L'altra questione, come abbiamo detto, è di merito: non si possono mettere assieme norme così eterogenee nello stesso decreto. Ma perché allora

che era stato presentato un programma di emendamenti e di ordini del giorno alla Camera, poi ripresentato al Senato. Ancora una volta, non avete voluto dare nessun segnale di lavoro comune

stiate andando a sbattere, perché avete deciso di imporre un modo di lavorare che prima o poi, chiaramente, porterà a dei risultati negativi, prima di tutto perché lo stiamo già vedendo dagli ultimi sondaggi: i giovani i giovani *under* 35 hanno dato dei segnali fortissimi nell'ultima campagna per le elezioni europee, non sono minimamente interessati alla vita politica per un motivo molto semplice, perché quando parliamo di questi temi loro non sono coinvolti in niente, questi temi non toccano le loro vite quotidiane, non c'è una relazione, non ci può essere una fiducia se non riprendiamo un lavoro parlamentare e non ci diamo delle regole ben precise su quello che deve fare un Governo e su quello che deve fare un Parlamento. Per tutte queste ragioni, il Gruppo Italia Viva voterà contro la fiducia.

Non so se sia un vero e proprio *record* quello che state raggiungendo, ma davvero siamo in una condizione francamente molto singolare, che penso vada stigmatizzata con forza in quest'Aula ancora una volta. Noi, come Alleanza Verdi e Sinistra, già alla Camera e naturalmente qui al Senato, con la presentazione dei nostri emendamenti, abbiamo cercato di evidenziare come questo decreto-legge accorpi - anche in questo caso non è certo la prima volta - argomenti, nel caso specifico, afferenti a quattro diversi Ministeri, una serie di norme frammentarie ed eterogenee (anche questo è stato detto) e nei nostri emendamenti, come spesso facciamo, abbiamo abbiamo cercato di migliorare questo testo, ma senza riuscirci, perché non sono stati presi in considerazione. Mi concentrerò ora, anche per esigenze di tempo, soltanto su una singola questione, quella dell'istruzione, che mi sembra particolarmente rilevante e che mi sembra anche riflettere appieno la visione e la cultura politica di questo Governo, che evidentemente è molto distante da noi. Questo provvedimento, infatti, dal nostro punto di vista, è pieno di insidie che impatteranno negativamente sul sistema formativo, sul sistema scolastico, aggravate per l'appunto da questa ormai rituale mancata accettazione delle proposte emendative e in questo caso anche della introduzione di nuove disposizioni peggiorative. Le misure relative al sostegno, al potenziamento linguistico per studenti che non conoscono adeguatamente la lingua italiana sono, a nostro avviso, particolarmente problematiche. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è riuscito a garantire un sistema di formazione e di reclutamento stabile e di qualità per l'inclusione degli studenti con disabilità, introducendo invece discrezionalità e discriminazione. Inoltre, le misure per il potenziamento linguistico sembrano davvero ispirate a logiche puramente escludenti. di mobilità aumentano il numero dei fuori sede; le modifiche alle procedure di valutazione dei dirigenti scolastici sono insoddisfacenti, trasformandosi in atti unilaterali del direttore del direttore generale. A questo si aggiunge che le ricercatrici ed i ricercatori sono condannati a una vera e propria di precariato permanente, senza tutele e senza diritti adeguati. Per garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2024-2025 sono previste risorse aggiuntive per il lavoro straordinario del personale del Ministero dell'istruzione e del merito finanziate tramite la riduzione del fondo di funzionamento destinato alle scuole; tuttavia, escludere il personale delle segreterie da questo riconoscimento è, a nostro avviso, profondamente ingiusto, soprattutto considerando che queste risorse aggiuntive saranno pagate direttamente dalle scuole. Il decreto-legge prevede, inoltre, la possibilità di stabilire nuovamente per decreto i criteri di riparto ed utilizzo delle risorse per il *tutor* e per l'orientatore, sottraendo queste prerogative alla contrattazione.

senza preavviso né motivazione gestionale, e assegna all'INDIRE compiti aggiuntivi legati alla formazione del personale scolastico; il testo prevede poi la sottrazione di 963 unità di personale ATA dalle scuole, che saranno messe a disposizione delle amministrazioni territoriali scolastiche senza possibilità di sostituzione. Come ben si capisce, questo provvedimento, coperto normativamente, esonera le amministrazioni da contestazioni contabili avanzate dal MEF. Sull'università, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane la giusta e grande preoccupazione dei rettori, che non crediamo si agitino a caso, perché il taglio al fondo di finanziamento ordinario rischia davvero di mettere in ginocchio i due terzi degli atenei. La questione del fondo di finanziamento ordinario è drammatica, molte università rischiano il *default*. Insomma, il decreto-legge rappresenta una serie di provvedimenti che, invece di migliorare il sistema scolastico, universitario e della ricerca, introducono ulteriori elementi problematici,

cento delle scuole ha una palestra; ci sono scuole che non hanno mense, non c'è il tempo pieno né il tempo prolungato, non ci sono strutture adeguate; abbiamo le famose - seppure una espressione che non amo - classi pollaio, abbiamo un mare di docenti precari. Sul terreno degli stipendi di questi insegnanti dobbiamo registrare anche in quest'Aula che, secondo secondo gli studi europei, nell'ultimo anno scolastico gli stipendi annuali degli insegnanti sono aumentati in una serie di Paesi per adeguarsi all'inflazione, ma non in Italia, dove invece sono diminuiti, per tutti i livelli di istruzione, dell'8 per cento. Questa, purtroppo, è la condizione di un Paese malato di diseguaglianza, in cui le istituzioni, lo Stato, che pure tutti noi rappresentiamo, non riesce a cambiare; una situazione in cui sempre di più e sempre più drammaticamente incidono la provenienza familiare, la diseguaglianza di origine sociale, le differenze nelle pratiche quotidiane, i divari nella qualità dell'occupazione dei genitori e degli studenti. Tutto questo alimenta la povertà educativa, distrugge il sogno delle pari opportunità e mina alla radice quel concetto di merito che avete ipocritamente voluto inserire nel nome del Ministero. Io ve l'ho detto già all'inizio di questa legislatura, ve l'abbiamo detto più volte: parlare di merito quando non sono assicurate le pari condizioni di partenza non solo è una grande ipocrisia,

a una logica egualitaria e si poneva esattamente il tema del superamento delle diseguaglianze. È insomma una spirale negativa che si trasmette inesorabilmente da una generazione all'altra, che segna il destino di tanti giovani, che mina le prospettive future anche economiche del nostro Paese. Una situazione che peraltro riflette davvero le profonde diseguaglianze educative presenti sul territorio nazionale le differenze tra il Meridione e il Nord del Paese. Di fronte a questa situazione che conosciamo, abbiamo in Aula un Governo che si presenta con questo tipo di provvedimento, peraltro qualche mese dopo - quindi in maniera da questo punto di vista davvero truffaldina

- cristallizza queste diseguaglianze e queste spaccature che esistono nel nostro Paese. Noi abbiamo chiesto tante volte, anche nell'esame qui al Senato, perlomeno di togliere perlomeno di togliere le norme generali dell'istruzione dall'autonomia differenziata, e questo invece purtroppo non è stato fatto. Capite bene che il combinato disposto di provvedimenti come questo e, dall'altra parte, l'autonomia danno proprio il senso di una visione che consideriamo profondamente sbagliata e che contrastiamo, perché da molto tempo a questa parte - e continuiamo ancora a farlo - ci battiamo invece per la dignità dei docenti e degli degli studenti. Per tutte queste ragioni, non smetteremo di contestare questo modo di fare che, dal nostro punto di vista, è completamente sbagliato.

Prima però la collega Sbrollini aveva richiamato all'attenzione l'interesse sui giovani. In realtà, una matrice unica e fondamentale in questo provvedimento c'è ed è proprio l'interesse politico di questo Governo nei confronti dei giovani, con un'attenzione particolare verso quelli più svantaggiati. Il filo conduttore è l'attenzione al benessere psicofisico e allo sviluppo dei giovani attraverso un approccio integrato che abbraccia sport, ricerca scientifica *housing* universitario e anche provvedimenti sull'istruzione e sulla scuola. Questi ambiti, che il collega giudicava distinti, sono in realtà interconnessi e fondamentali per creare un ambiente stimolante e sostenibile per i nostri giovani. Le misure introdotte mirano a creare opportunità concrete, permettendo ai giovani di esprimere il proprio potenziale e di contribuire attivamente allo sviluppo della società. Il supporto agli studenti universitari, il miglioramento delle condizioni di lavoro per i giovani ricercatori, la promozione della pratica sportiva sono tutti tasselli di una strategia molto più ampia che aiuta a costruire una società più equa e dinamica. Lo sport, con le sue regole di trasparenza e di *fair play*, insegna ai giovani i valori essenziali come la disciplina, la perseveranza e il rispetto delle regole. Questi stessi valori li ritroviamo nella ricerca scientifica, dove l'integrità e la trasparenza sono alla base del Allo stesso modo anche garantire affitti equi per gli studenti universitari non è solo una questione economica, ma un modo di assicurare che tutti i giovani abbiano le stesse opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione. In questa ottica, il Governo riconosce che investire nei giovani significa non solo fornire le risorse necessarie, ma anche creare un ambiente dove possano crescere, imparare e contribuire attivamente alla società. Le misure introdotte sono pensate per sostenere i giovani in tutti gli aspetti della loro vita, dal campo sportivo al laboratorio di ricerca, fino alla loro vita quotidiana come studenti universitari. Riguardo allo sport è giusto che la politica se ne interessi, ma solo per salvaguardarne la necessaria autonomia e garantire la trasparenza delle fondazioni e degli enti sportivi. mirano a rafforzare la fiducia nelle istituzioni sportive attraverso la regolamentazione e la semplificazione burocratica, rendendo più accessibile la pratica sportiva a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche. La valorizzazione del lavoro sportivo volontario e la regolazione dei compensi sono passi essenziali per assicurare che tutti coloro che contribuiscono al mondo dello sport siano riconosciuti e sostenuti adeguatamente. Si rischiava altrimenti di perdere figure considerate amatoriali, ma fondamentali per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica (chi prepara la gara, per esempio, e chi è ufficiale di gara). Poi c'è l'intero capo del provvedimento dedicato al sostegno della ricerca e delle università. Grazie al ministro Annamaria Bernini, c'è innanzitutto la proroga per consentire la riforma dei contratti di ricerca. Sappiamo quanto sia delicato il campo della ricerca e quanto i giovani laureati siano attratti da altre realtà nel mondo. Riuscire ad attivare ulteriori strumenti contrattuali per attrarre nel sistema della ricerca universitaria giovani di talento diventa fondamentale, prevedendo strumenti efficaci e flessibili, a tutela crescente, accompagnati dalle necessarie coperture finanziarie. Così come, grazie a una norma di questo provvedimento, ci sono le risorse economiche per l'assunzione dei ricercatori universitari in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in qualità di professori universitari di seconda fascia. Inoltre, grazie a un emendamento dei nostri colleghi alla Camera, è stato più che raddoppiato il fondo destinato ai contributi agli studenti universitari che devono provvedere ad affitti fuori sede, al di fuori degli studentati. La riforma dell'*housing* universitario, legata ai fondi del PNRR, è in fase di realizzazione e questa misura si muove proprio nel senso di accompagnarla, sostenendo gli studenti in un momento in cui il caro degli affitti sta diventando pesante per alcune famiglie. È stata inserita anche una misura per garantire il diritto allo studio degli studenti con gravi disabilità, prevedendo appunto degli assegni a favore del personale specializzato che assiste lo studente durante le lezioni universitarie. Il settore dell'università e della ricerca è vitale per il progresso e la competitività del nostro Paese. Grazie a questo provvedimento e grazie al ministro Bernini si introducono misure che offrono maggiore flessibilità e supporto ai giovani ricercatori sostegno economico agli studenti universitari, in particolare a quelli fuori sede, che hanno condizioni sfavorevoli. Questo serve per attrarre e mantenere i talenti, per evitare la fuga dei cervelli e per promuovere l'eccellenza accademica. C'è poi un vasto pacchetto di misure volto a garantire l'avvio dell'anno scolastico, che partirà a settembre e che riguarda il personale docente, quello amministrativo e quello ausiliario. Viene prevista la fornitura gratuita dei libri di testo per gli studenti meritevoli che abbiano determinati requisiti, così come sono anche previste una serie di disposizioni per tutelare il diritto degli alunni con disabilità. L'attenzione è rivolta in particolare al profilo professionale del docente specializzato nel sostenere gli alunni disabili. Per tutte queste ragioni, il Gruppo Forza Italia esprime un voto favorevole. Siamo convinti che queste misure non solo rispondano alle urgenze immediate, ma pongano anche le basi per un futuro più inclusivo e competitivo per il nostro Paese. garantire la trasparenza nelle attività sportive e supportare la ricerca scientifica sono elementi chiave, tutti insieme, per costruire un'Italia migliore e capace di affrontare le sfide del futuro.

elemento fondamentale e fondante di chi fa sport, di chi va a scuola e di chi frequenta l'università: l'esercizio alla democrazia, allo stare insieme, al confronto, anche alla sana rivalità e al sano scontro. Solo che questo esercizio democratico che si fa nello sport, a scuola e all'università qui oggi è negato. Oggi, in maniera plastica in la democrazia è stata bocciata. Sì, perché in Commissione non è intervenuto nessuno della maggioranza e non ho avuto il piacere di sentire le argomentazioni Oggi in discussione generale è intervenuta essenzialmente l'opposizione e, forse per educazione, c'è stato l'intervento di un esponente di Fratelli d'Italia. Questa è democrazia? Come si fa a parlare di un tema fondamentale come la scuola e di altri temi importanti importanti come lo sport e l'università in quarantott'ore? Non penso che la scuola meriti questo. E poi, permettetemelo: abbiamo presentato poco più di 100 emendamenti che penso davvero potessero anche essere affrontati

non parlare mai di scuola. Doveva essere la prima donna Presidente del Consiglio a non parlare quasi mai di scuola, e dico quasi mai perché può essermi sfuggito qualche intervento. *(Applausi)*. Di armi sì, ma di penne, matite e libri mai, tant'è vero che è stato importantissimo chiedere lo scorporamento degli investimenti in armi, mica quelli in istruzione. Ovviamente ognuno ha le sue priorità: mi chiedo dove sia la collega che nella scorsa legislatura tanto si batteva il petto sulla scuola e che adesso è silente e fa solo qualche intervento in dichiarazione di voto e nulla più. Parliamo però di soldi e risorse, perché può anche non parlarne un Presidente del Consiglio. Vedete, tutti i Ministri dell'istruzione chiedono soldi. Chi è il Ministro che non chiede soldi per il proprio Ministero? Sarebbe sciocco, no? E non ho dubbi che il ministro Valditara abbia chiesto risorse per la scuola. La differenza sapete chi la fa? E lo sapete meglio di me, perché me lo insegnate, visto che da una vita siete qua dentro, mentre io Presidente del Consiglio che orienta all'incirca e, quindi, agevola. Ed è con Conte presidente del Consiglio che sono stati stanziati 10 miliardi per la scuola, non con Giorgia Meloni. *(Applausi)*. Noi in questo provvedimento cos'abbiamo? 500 milioni di risorse fresche, perché le altre già esistevano e vengono spostate da qua a là, cambiano nome, ma sempre sono quelle, poche e minime. L'avrei

tra i Ministri della Lega: prima infatti c'è Salvini per il Ponte e quei 16 miliardi servono lì, meglio un ponte di cultura che un ponte di cemento, a parer mio. E poi chi

possa non valere tanto quanto quello di un ragazzo che si diploma in un'altra Regione. Il ministro Valditara, quindi, è l'ultimo degli ultimi anche all'interno del proprio partito. Secondo me, invece, dovrebbe combattere per la scuola. Giorgia Meloni non gli dà le risorse, almeno all'interno del suo partito non si faccia mettere proprio all'ultima fila, perché sarebbe veramente un peccato. Perché questa sessantesima fiducia? Non certo perché noi abbiamo fatto ostruzionismo. Posso essere un po' piccata, possiamo anche criticare; abbiamo presentato anche emendamenti che ritengo vagamente di buonsenso; mi permetterete l'arroganza di poter dire che possiamo aver scritto qualcosa anche di intelligente e accoglibile, che invece è stata

E cosa tiene insieme questo decreto-legge? Certamente le motivazioni nobili che ha detto il senatore Occhiuto e quelle che ho aggiunto io sul valore democratico di grandi temi quali sport, scuola e università, ma soprattutto due l'occupazione. Per voi è importante e io vi do ragione. Infatti in questo provvedimento c'è l'occupazione dei posti di potere e lo state facendo sia per lo sport che commissariando l'INDIRE; *spoils system,* altre poltrone. È così, è un dato di fatto. Tutti i bei termini nobili che lei ha usato, collega, in questo provvedimento non ci sono. Ci sono posti e nomine da

discriminazione, perché voi discriminate chi è professore e insegnante di sostegno che ha fatto un percorso da altri che potrebbero farne un altro; chi ha vinto un concorso da dirigente

Decide di portare in dono dei capponi e li tiene per le zampe. Sono ancora vivi e quei capponi, scossi dall'agitazione di Renzo che cammina e che si immagina cosa dirà mai all'Azzeccagarbugli, vengono sbattuti gli uni contro gli altri, altri, e, andando tristemente verso lo stesso destino - quello della cucina, il destino di essere uccisi e mangiati - beccano tra di loro. Ecco quello che andate a fare con questo provvedimento. Continuate a mettere gli uni contro gli altri di uno stesso sistema che invece andrebbe armonizzato.

con questo provvedimento vengono introdotte misure significative che segnano un ulteriore passo in avanti nell'azione riformatrice del Governo in tema di sport, scuola e università, soprattutto con interventi per il sostegno didattico agli studenti con disabilità. In tema di sport, come Lega riteniamo che i provvedimenti presi da questo decreto-legge vadano nella giusta direzione, anzi di più: siano funzionali a quella grande operazione di radicale rinnovamento di cui necessita in particolare il nostro calcio. Serve infatti riformare le fondamenta dell'intero movimento calcistico italiano con un grande piano di sviluppo del talento, con la programmazione, l'organizzazione e soprattutto nuovi impianti sportivi. A problemi strutturali servono soluzioni strutturali, nuove idee e soprattutto nuovi interpreti. Sono passati ormai dieci anni dall'ultima partita della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali e uscire in quel modo dagli Europei, soprattutto dopo due mancate qualificazioni ai Mondiali, è l'ennesima vergogna sportiva che gli italiani non meritano. C'è modo e modo di perdere e c'è modo e modo di assumersene la responsabilità. Questo tracollo sportivo, comunque, parte da lontano. Do alcuni numeri per analizzare la situazione. Basti pensare che nella Liga spagnola giocano 435 giocatori spagnoli; in Bundesliga giocano 362 giocatori tedeschi; in Serie A, ormai, sono meno di 300 gli italiani che, oltre ad essere poco impiegati in Italia, sono quasi totalmente assenti negli altri grandi campionati europei. Si pensi che nelle quattro massime serie di Inghilterra, Spagna, Germania e Francia i giocatori italiani sono in tutto solo una ventina. Inoltre, gli sconti fiscali del decreto crescita hanno aiutato inizialmente i conti in rosso delle nostre società, ma, a lungo termine, hanno agevolato acquisti di giocatori stranieri dall'estero. Tutto a danno dei talenti italiani e a farne le spese è la Nazionale. Bene ha fatto il ministro Salvini ad opporsi e a bloccare l'ennesima proroga, introducendo invece il grande tema delle infrastrutture e dei nuovi stadi. Per quanto riguarda il decreto-legge in oggetto, quindi, è giusto intervenire sul tema della rappresentanza per le Leghe professionistiche, anche in virtù del contributo economico apportato al sistema sportivo. Giusto riformare il sistema dei controlli, introducendo una commissione che svolga l'attività di vigilanza sulla regolarità Veniamo alla scuola. Per quanto riguarda gli interventi sulla scuola, sono previste misure che riaffermano in maniera più incisiva l'importanza di un sistema educativo che prenda davvero in carico gli studenti più fragili, in particolare gli studenti con disabilità. Con questo spirito, quindi, sono previste alcune misure per tutelare il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti con disabilità. Servono innanzitutto docenti sempre più competenti e motivati, ma soprattutto serve che il sistema sia in grado di garantire docenti specializzati sul sostegno didattico Pertanto, bene ha fatto il ministro Valditara a intervenire alla radice del problema, caratterizzato, da un lato, dalla grave carenza di docenti specializzati sul sostegno

Finora nessuno si era fatto carico del problema, che pure era sotto gli occhi di tutti. A fronte di un'offerta formativa universitaria fortemente diseguale sul territorio, si assisteva infatti al al susseguirsi di supplenze dei docenti di sostegno, che impediva loro, di fatto, come in un circolo vizioso, anche di seguire i corsi di specializzazione. Inoltre, è del tutto evidente che i docenti precari, che svolgono già da anni e con merito l'attività di insegnamento sul sostegno, abbiano bisogno di percorsi formativi con contenuti mirati e differenziati rispetto ai corsi universitari che sono rivolti indistintamente anche a giovani neolaureati senza esperienza di insegnamento. Questi nuovi percorsi saranno di qualità e innovativi e coinvolgeranno il mondo delle associazioni delle persone con disabilità. È stata poi introdotta un'altra importante iniziativa, che mira a porre un argine al mutamento continuo dei docenti supplenti, davvero non più accettabile. Mi riferisco alla possibilità di ottenere la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico su richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità, previa valutazione da parte del dirigente scolastico e dell'interesse dell'alunno, affinché il rapporto virtuoso tra docente e studente non si interrompa. Con questa misura si rafforza il rapporto tra la scuola e la famiglia, soprattutto in un ambito dove questo rapporto deve essere necessariamente stretto. con questo decreto viene affrontato un altro annoso problema, quello del contenzioso su titoli esteri dei docenti con abilitazione all'estero, distinguendo tra i titoli acquisiti presso atenei seri e accreditati e quelli acquisiti presso enti inaffidabili. Con le nuove disposizioni si supera il tema oggetto di contenzioso per offrire ai circa 11.000 soggetti con istanza di riconoscimento pendente di poter accedere a percorsi di specializzazione *ad hoc*. Abbiamo, infine, introdotto una misura doverosa per gli studenti di origini straniere che, in particolare se appena arrivati in Italia, non possiedono un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana. Le nuove misure consentono loro di acquisire una conoscenza adeguata dell'italiano mediante corsi dedicati di potenziamento linguistico. La competenza linguistica dell'italiano è requisito fondamentale per un'integrazione che sia vera e non solo predicata, perché non si integrano gli alunni stranieri oscurando le nostre radici culturali, togliendo i crocifissi dalle scuole, vietando i canti di Natale o sospendendo le lezioni per il Ramadan: si integrano insegnando *in primis* la lingua italiana, la nostra cultura e i nostri valori. In questo modo anche i bambini stranieri potranno godere di quell'ascensore sociale che può essere la scuola. Anche sull'università si va nella giusta direzione. Penso alle misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con gravissima disabilità e all'incremento di 10 milioni di euro del fondo per dare un contributo per le spese di locazione abitativa agli studenti che hanno un ISEE familiare non superiore ai 20.000 euro. È per tutto questo, per quanto ho sinteticamente per quanto ho sinteticamente illustrato, che questo decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'azione riformatrice del Governo e perciò annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega.

Siamo forse a 70, con 59 fiducie, di cui 23 in Senato, e in questo sistema di monocameralismo alternato - come ha ricordato la senatrice Malpezzi - noi al Senato praticamente non abbiamo potuto discutere

al tetto della spesa per i libri di testo, adeguandola all'inflazione: misura richiesta perché oggettivamente il materiale costa di più, ma che oggettivamente comporterà un aumento della spesa da parte delle famiglie, il decreto prevede solo 3 milioni in più per il sostegno alla spesa dei libri per la scuola dell'obbligo. Come ricordava stamattina sempre la senatrice Malpezzi, solo per la scuola dell'obbligo, il fabbisogno

muoversi rispetto a quelli che occuperanno solo per un periodo il posto che non sono riusciti a occupare quelli che faranno il concorso, che in molti luoghi non è ancora finito.

norme che riguardano l'inizio dell'anno scolastico, andrebbe dato modo ai due rami del Parlamento - e quindi anche a questo - di intervenire su norme che vengono richieste anche su emergenze che si pongono, come quella di dare il tempo e fare una proroga per l'iscrizione all'albo degli educatori degli educatori dei Comuni; norme, quindi, che sono state cambiate in Aula alla Camera, che si aggiungono a quelle che il decreto-legge già conteneva e che non ci hanno convinto: alla riforma della modalità di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali delle discipline associate e degli enti di promozione che compongono il CONI e il Comitato paralimpico. Salta il limite ai mandati, ma noi abbiamo soprattutto posto il tema della questione dei metodi: la parità di genere, l'accesso ai giovani, il voto elettronico; cose che abbiamo cercato e riproposto in un ordine del giorno che, molto riformulato e molto edulcorato, stamattina

se la crisi del calcio è un tema di identità nazionale, rispetto al fatto che le altre squadre hanno tanti giocatori nazionali. Io so che le altre nazionali hanno tanti giocatori di un popolo plurale in in cui riconoscono i nuovi cittadini, mentre noi fatichiamo tantissimo a riconoscere i nuovi cittadini. *(Applausi)*. Poi c'è la scuola: i titoli sono buoni, si parla dell'inclusione, però lo svolgimento è totalmente sbagliato. Anche su questo noi avremmo voluto dare una mano e anche su questo si creano percorsi paralleli. La senatrice Barbara Floridia, citando Manzoni, ha parlato dei capponi che si beccano. un pasticcio: percorsi paralleli temporanei, tra l'altro affidati a INDIRE, che creano disparità di trattamento e abbassano la qualità della formazione, con l'idea che la formazione seria e qualificata di sostegno organizzata dagli atenei ha un valore secondario di fronte all'emergenza e a criticità croniche, che andrebbero affrontate con risposte strutturali, a cominciare dagli organici. Mi dispiace dire al senatore Paganella, tramite lei, signor Presidente, che non è vero che è la prima volta: se sono potuti entrare circa 25.000 docenti di sostegno, è perché ci sono state manovre di altri Governi.

posti vacanti e precari. Però questa questione va affrontata senza abbassare il livello di formazione, perché la continuità è prima di tutto un diritto di quegli studenti, non è un bisogno *à la carte* delle famiglie. È un diritto dei bambini e e delle bambine e lo si garantisce con l'organico e uscendo dalla precarietà. In questo caso, invece, siamo di fronte a scorciatoie che umiliano chi ha studiato. A queste criticità, si aggiungono quelle del Servizio sanitario nazionale che voi non finanziate, con i ritardi sulle diagnosi che hanno bisogno di tempo e di *équipe*. Quei bambini e quelle bambine hanno bisogno di un *welfare* che funziona. Il provvedimento inserisce - ed è un tema molto delicato e serio - la possibilità di creare percorsi di conferma su richiesta delle famiglie. È un tema serissimo e qui il Ministro ci ha ricordato l'articolo 30 della Costituzione: è dovere dei genitori sostenere, mantenere, istruire ed educare i figli. Certo, è dovere dei genitori ed è una loro responsabilità e l'educazione è qualcosa di complesso che riguarda la persona nei suoi vari ambiti, però i genitori non sono insegnanti. Poi ci sono le competenze, che si acquistano nella scuola, e c'è l'articolo 34, secondo il quale la scuola è aperta a tutti e la Repubblica rende effettivo il diritto allo studio. Il tema del diritto allo studio dei bambini con disabilità non si può risolvere con la richiesta della singola famiglia, perché l'insegnante agisce in un gruppo-classe, collabora a un progetto educativo. È un problema di didattica serissimo; un progetto educativo che fa maturare al massimo le potenzialità dei ragazzi e delle ragazze. I nostri emendamenti andavano in un senso che rafforzava la verifica di quel processo di inclusione approvato dal gruppo di lavoro sull'inclusione. L'insegnante di sostegno lavora non solo sul singolo, ma sul gruppo-classe, perché sostiene tutti. Il tema è creare un ambiente che sostiene il bambino o la bambina con degli altri bisogni. Mi soffermo poi su INDIRE, a cui abbiamo affidato questi percorsi, che viene commissariata. Diamo nuovi incarichi e ampliamo,

lavorare sull'italiano - e non sono solo questi i bisogni - in modo separato fuori, dalle ore di curricolo: è riduttivo questo modo ed è a rischio di segregazione. Voglio ricordare - perché questo è il tema del decreto-legge - che, tra la produzione di norme e la realtà, c'è lo spazio di governo dei fenomeni sociali, ci sono le pratiche sociali, c'è la comunità educante, c'è il terzo settore, ci sono le buone pratiche che questo Governo non vede mai quando interviene

se proroga ulteriormente la riforma che superava l'assegno di ricerca, che è il simbolo della precarietà giovanile nell'università? Dodici anni nel pre-ruolo.

di precariato nell'università. Come si fa a dire che si supera una riforma, che non si è voluta attuare e prima ancora di attuarla - una riforma pensata nella crisi del Covid e legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza - mentre si taglia il fondo di funzionamento ordinario delle università statali e quei soldi per i ricercatori entrano in quel fondo? C'è un allarme che i rettori hanno dato, e mai in questo modo: la CRUI non è un comitato di pericolosi rivoluzionari; mai in questo modo un allarme così grande era stato lanciato dai rettori, per un fondo che riguarda il funzionamento del sistema. Il dubbio che ci viene è che si pensi che alla grande massa ci pensano le telematiche, magari neanche quelle di qualità, e che poi ci sono le università private e il resto, il sistema pubblico, può anche deteriorarsi. Noi siamo contro questa ipotesi, voteremo contro questa fiducia e siamo contro la politica che questo decreto-legge

prima di entrare nel merito del provvedimento, desidero rispondere, tramite la sua persona, alla senatrice Floridia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è abituato a perdere tempo, non è abituato a fare non è abituato a *spot* pubblicitari o, peggio ancora, non è abituato a fare provvedimenti già famosi per avere distrutto il nostro tessuto economico. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa fatti con questo decreto, che è anche uno dei tanti che dimostra che è il Governo del fare, è il Governo che pensa di creare un futuro per le nuove generazioni. Inoltre, tengo a precisare che la senatrice stamattina ha avuto tutto il tempo necessario per potere grazie alla gestione da parte del presidente Marti, che ringrazio. Ha avuto tutto il tempo per chiarire e per dimostrare il suo pensiero sugli emendamenti e sugli ordini del giorno. Ma non solo: ha avuto le risposte che ha chiesto da parte del Ministro, visto che il Ministro era presente stamattina in Commissione. Quindi, non capisco le sue lamentele o, meglio, le capisco, perché il MoVimento 5 Stelle sa solo dire falsità e bugie e continua a negare i *(Applausi)*. Forse la senatrice, per la sua rarissima presenza in Commissione, voleva un tappeto rosso. al decreto. Questo - come ho già detto - dimostra la grande attenzione, da parte del Governo Meloni, su settori strategici e fondamentali, come lo sport, il sostegno agli alunni con disabilità, l'università e la ricerca. Grazie al lavoro dei Ministri di competenza, che ringrazio, sono state introdotte tante misure importanti, che riguardano la vita dei nostri giovani e soprattutto dei più fragili. È proprio sui più fragili che voglio soffermarmi. Grazie che accresce effettivamente il supporto agli studenti più fragili. Negli ultimi anni, infatti, a causa della poca attenzione riservata da parte dei precedenti Ministri al tema della tutela degli studenti con disabilità, nonostante i

per assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati. E ciò è dovuto anche al fatto che l'offerta formativa universitaria in tutti questi anni non è riuscita ad allinearsi al fabbisogno, anche perché c'è stata una grande grande disomogeneità in termini di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Tutto ciò cosa ha determinato? Ha determinato che oggi siamo in una situazione veramente drammatica. Abbiamo 85.000 docenti privi di specializzazione sul sostegno e 136.000 alunni che non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati. E voi opposizione dite che non era necessario intervenire subito, che non era una materia urgente su cui intervenire subito? Ringrazio invece il ministro Valditara, che ha capito quanto fosse necessario e urgente affrontare subito e risolvere la criticità connessa alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno e rafforzare così l'azione l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili. E quindi cosa si è fatto? Si è previsto un potenziamento dei percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa. Infatti, la specializzazione nel sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita anche mediante il superamento di percorsi che saranno attivati dall'INDIRE, nuovi percorsi di formazione con contenuti innovativi e soprattutto mirati alle reali esigenze formative di questi docenti, lo ricordo, sono rivolti a una platea ben definita, i triennalisti, che già operano attraverso le supplenze in forza delle quali oggi hanno un'esperienza di fatto, anche se privi di specializzazione nel sostegno. Ancora una volta, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alle opposizioni: è inutile, smettetela di gridare allo scandalo e dire che c'è una disparità di trattamento tra docenti o sanatorie. Questa misura ha l'obiettivo di ridurre in modo considerevole la platea dei precari triennalisti, che siete bravi a scendere nelle piazze e battere il petto per difendere, per poi andare contro un reale provvedimento che ha l'obiettivo

che stabilirà i nuovi contenuti vedrà per la prima volta il coinvolgimento dell'osservatorio per l'inclusione scolastica in modo da dare veramente una formazione attraverso il suo contributo con percorsi più innovativi e ambiziosi. Si risolve anche l'altra annosa questione delle istanze giacenti per il riconoscimento dei titoli esteri. Tengo a precisare che questa situazione non è nuova, ma l'abbiamo

pur garantendo un livello formativo adeguato per coloro che conseguiranno la specializzazione nel sostegno. Si tratta di 11.000 docenti che, proprio per la carenza formativa universitaria, non sono riusciti a prendere la specializzazione, quindi sono stati costretti, nel tempo, a prendere l'abilitazione in uno o più Stati membri dell'Unione europea. Inoltre,

alle normative europee, perché l'Europa non è qualcosa che diciamo che ci piace e dove vogliamo andare, ma poi, quando non ci conviene, non vanno bene le norme europee. Abbiamo fatto di più, però: attraverso questi percorsi formativi, diamo una maggiore formazione, perché sappiamo quanto sia importante e delicata la funzione del docente di sostegno. Infine, parlate tanto di garantire la continuità didattica per i nostri alunni e anche questa volta, allo scandalo: la famiglia non entra nelle scuole, ma entrano gli estranei nelle scuole. Bene: in queste Aule, in questi giorni, nei vari dibattiti abbiamo detto che dobbiamo intensificare il rapporto che c'è tra

Nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno, i docenti che sono stati in servizio su un posto di sostegno nell'anno precedente e che rientrano nel numero dei nominandi

per la serenità di questi ragazzi con disabilità. Lo abbiamo fatto - vivaddio - e voi gridate allo scandalo dicendo che la famiglia non deve entrare nella scuola. In sintesi

Sono state emanate misure per il funzionamento degli organismi sportivi, in particolare in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali. Si tratta sicuramente di misure necessarie. Sono state previste altresì norme in materia di prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici coinvolti in attività sportive e in materia di rimborsi forfettari per i volontari sportivi. Tali cambiamenti semplificano la materia e riducono la burocrazia, favorendo una maggiore flessibilità. In sintesi, Presidente, Presidente, questo provvedimento si incardina perfettamente in quel sistema di riforme che il Governo Meloni porta avanti sin dal suo insediamento che dimostra, come ho già detto e voglio ancora una volta ribadire, quanto questo Governo sia il Governo del

in 6a. Oggi sono passata in quella Commissione per seguire. La presenza in quest'Aula non è uno scherzo e non dico inesattezze o falsità. Per me questo è un luogo sacro. Per me.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

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore

votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1193, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, nel testo approvato dalla Camera dei deputati,

io ho bisogno di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla vicenda di Trenitalia che, dal 22 al 26 luglio, ha sostanzialmente sospeso il trasporto ferroviario passeggeri nelle linee da Sapri in su,

Sud. Persone che avevano prenotato il viaggio per potersi recare a fare concorsi, per fare adempimenti importanti, si vedono recapitare un messaggio da Trenitalia con il quale vengono invitati a trovare un modo un modo alternativo per raggiungere la destinazione con l'avviso che il rimborso del titolo di viaggio sarà fatto entro un anno dalla data della richiesta. Io ritengo che Trenitalia non si possa permettere di sospendere e di cancellare e di cancellare per cinque giorni la gran parte dei viaggi e dei treni che partono da Sapri verso le destinazioni del Nord Italia, perché questa è una ulteriore dimostrazione di come questa Italia sia a due velocità. Signor Presidente, le chiedo di farsi portavoce di questa mia lamentazione vera e propria con il ministro Salvini, perché ritengo che nel 2024 un disservizio tale non sia francamente degno di uno Stato moderno e certamente non di un Governo che dice di voler realizzare il Ponte sullo Stretto, che dovrebbe avere la linea ferroviaria, oltre che quella autostradale, e poi per cinque giorni taglia fuori il Sud dal trasporto ferroviario.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo oggi in quest'Aula per portare alla vostra attenzione un fatto gravissimo e di una violenza inaudita che si è verificato giovedì nel carcere di Salerno, nella casa circondariale di Fuorni. Un detenuto ventiquattrenne ha aggredito con una lametta da barba il suo compagno di cella trentenne, del quale pare tra l'altro si occupasse perché quest'ultimo non era in grado di deambulare autonomamente. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento da parte della Polizia penitenziaria, l'aggredito è successivamente deceduto all'ospedale Luigi d'Aragona. Signor Presidente, una cosa mi preoccupa più di altre ed è un pensiero ricorrente in questi giorni in cui, in Commissione giustizia, di cui faccio parte, stiamo esaminando il decreto carceri al centro del dibattito parlamentare e non. La mia paura, signor Presidente, è che, con l'aumento di questi episodi gravissimi, possa radicarsi il pensiero pericolosissimo che tutto questo sia normale, quando è inaccettabile. Come è inaccettabile che nel carcere di Salerno ci siano 572 detenuti in luogo dei 372 che la struttura può ospitare. È inaccettabile che gli agenti in servizio siano 128 e debbano fare il lavoro che dovrebbero fare in 243. Presidente, un'altra cosa per me è inaccettabile, e mi rivolgo per il suo tramite ai colleghi di maggioranza. È questo disco rotto che l'emergenza non l'ha creata il Governo; che questa maggioranza non è responsabile di quello che sta succedendo. Ricordo prima a me stessa, evitando di andare in confusione, essendo io avvocato, che questo non è un tribunale. Qui dentro non facciamo processi, ma cerchiamo di trovare delle soluzioni per quello che succede fuori. allora: quale soluzione vogliamo trovare, se nel decreto carceri che stiamo analizzando è stato previsto uno stanziamento di mille assunzioni straordinarie, mentre quelli che ci sono stati prima, da cui spesso i colleghi di maggioranza sembrano essere ossessionati, di assunzioni, con un tale Bonafede, ne hanno fatte 4.000, straordinarie e finanziate? Presidente, una materia così delicata non può essere trattata sull'onda emotiva di fatti di attualità, nemmeno possiamo permetterci, come recita un noto detto partenopeo, che mentre il medico studia, il malato muoia. Pesano sulle nostre coscienze delle responsabilità grandissime ed è tempo di abbandonare atteggiamenti giustificazionisti ed onorarle. Ha ragione, è un tema molto delicato, difficile da affrontare anche in un intervento di fine seduta. interviene su un anniversario importante.

69 adolescenti, ragazzine e ragazzini giovanissimi che partecipavano a un campeggio organizzato dai socialisti e laburisti di quel Paese. Lo fece con barbara ferocia e lucidità, per odio contro l'Europa, i migranti, il multiculturalismo, la società aperta. Un crimine e una strage che scossero il mondo intero, in nome di farneticazioni razziste, suprematiste e neonaziste tredici anni fa, non fa, quando il nazismo le stragi le pianificava con il genocidio pianificato della Shoah, con i campi nei quali vennero sterminati milioni di ebrei, omosessuali, disabili, rom, comunisti e antifascisti. Posizioni che Breivik mantiene ancora oggi dal carcere dove si trova e dove comunica molto con l'esterno, con esternazioni deliranti e pericolose, con proclami a favore delle destre estreme che operano in Europa e nel mondo, posizioni contro l'ONU, contro la NATO, contro l'Europa, a favore di Putin Putin e anche di Trump, quello di Capitol Hill, contro il dialogo euro-arabo e interreligioso, su posizioni islamofobiche. Questo in un mondo che rischia di esplodere, dove in questi anni, in questi mesi dilagano anche antisemitismo, odio e dove altre stragi dello stesso segno scandiscono questo tempo. con un altro pensiero: noi vogliamo ricordare ancora oggi quella strage e quei pericoli. Nessuno può girarsi dall'altra parte, anche nel nostro Paese. È ancora viva l'emozione che provammo cinque anni fa, quando a Macerata un estremista di destra sparò per le strade ferendo sei immigrati. Simili le motivazioni, stesso l'odio. Vogliamo cogliere questa occasione e questo momento per citare un episodio di soli tre giorni fa che si inserisce in queste scie di odio e di rigurgiti dell'estremismo. Mandiamo allora un abbraccio e una forte solidarietà ad Andrea Joly, giornalista della «Stampa» aggredito con violenza a Torino da militanti di CasaPound mentre riprendeva i loro gesti e le loro manifestazioni ispirate a un neofascismo. È molto importante che la condanna di quell'episodio sia stata generale, come si dice multipartisan, ma pensiamo - Presidente, le chiedo se può anche trasferire questa nostra

Parlo dei tempi, non dei temi.